finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da* handicap *in situazione di gravità*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato

con il seguente testo: «Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5». Cosa si diceva? La Commissione

soppresso questo articolo di buonsenso. Noi, come Gruppo, avevamo dato il nostro parere favorevole ed avevamo votato favorevolmente questo disegno di legge, proprio perché andava verso le garanzie costituzionali. No!

il Presidente del Senato e non capisco perché non lo faccia - non esistiamo più. Altro che la soppressione costituzionale! Ci hanno già soppresso, perché la nostra volontà viene sempre respinta politicamente. Qui andiamo avanti solamente per aumentare le pene, niente di più e niente di meno.

non è neanche "populista", perché sulla giustizia il popolo la pensa come vi sto dicendo io. Il popolo, infatti, dice che una gamba va

È questa la tortura ed è qui che ogni anno dalla Corte europea di giustizia subiamo condanne e paghiamo. Tutte le professioni pagano sulla responsabilità civile, tranne una, quella degli

che ci sono state date dai nostri Padri costituenti.

- un no chiaro e forte, perché non vogliamo essere coinvolti. Prima o poi, infatti, il popolo dovrà fare veramente quella rivoluzione socialista che aspettiamo ed i giustizialisti dovranno essere cacciati

interviene in maniera efficace sul punto che intendeva trattare, rendendo più strette le maglie del ricorso alla custodia cautelare.

aver sottoposto un gruppo di suoi cittadini ad un episodio violentissimo e gravissimo di tortura, sta cercando a venirne fuori, mettendo in campo i rimedi per una sanzione applicata già più di due anni fa, e anche in quel caso per aver sottoposto una fascia di cittadini ad un trattamento inumano e degradante. Mi riferisco alle persone ristrette all'interno di istituti di detenzione in una situazione di sovraffollamento eccessivo rispetto ai minimi *standard* previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani. Oggi stiamo uscendo da quella situazione:

che poi salgono a 122 se consideriamo i posti in istituti carcerari che oggi non sono disponibili a causa di lavori di ristrutturazione. Parliamo, cioè, di una popolazione complessiva di 54.000 detenuti, a fronte di una capienza di quasi 50.000 posti. Siamo ancora in una situazione di sovraffollamento, ma abbiamo 8.000 detenuti in meno rispetto al gennaio del 2013.

Tra i tanti punti ancora oscuri, ne rimane però uno ancora molto grave, ovvero la percentuale dei ristretti nelle nostre carceri in stato di custodia cautelare. Se andiamo a vedere quel dato, siamo ancora del tutto fuori dalla media europea.

in stato di custodia cautelare o con sentenza non definitiva, a fronte di una media europea del 21,5 per cento. È questa una delle situazioni che necessita un più urgente intervento. Il disegno di legge in esame, che mi auguro venga oggi approvato definitivamente, va per l'appunto nella direzione giusta. Esso va intanto nella direzione di limitare la discrezionalità del giudice nell' applicazione della custodia cautelare, limitando i casi in cui il pericolo di fuga o la situazione di possibile reiterazione del reato possano essere utilizzati come motivazioni per la custodia cautelare. Si inserisce, quindi, l'elemento dell'attualità accanto a quello della concretezza, per definire la pericolosità o meno del detenuto, rispetto al pericolo di fuga o di reiterazione del reato, e si prevede che non possa essere il titolo del reato in sé a definire il pericolo di fuga o di reiterazione

3 - secondo cui non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere, se il giudice ritenga che, con sentenza finale, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2014, sui risarcimenti ai detenuti e le modifiche dell'ordinamento penitenziario, in cui abbiamo stabilito che il giudice non può applicare la misura della custodia cautelare in carcere se ritiene che, all'esito della pena, la detenzione non sarà superiore a tre anni. Si ha, quindi, un margine più ampio rispetto al limite dei due anni sotto il quale è concessa la sospensione condizionale della pena. Non c'è stato, pertanto, alcun passo indietro, neanche su questo punto. Abbiamo Abbiamo inoltre previsto che l'obbligo di custodia cautelare in carcere venga definito solamente per alcuni gravissimi reati, ovvero l'associazione sovversiva, l'associazione terroristica e l'associazione mafiosa. Sono rimasti fuori da questo obbligo altri reati pure molto gravi: penso - ad esempio - a tutti i reati relativi al maltrattamento dei minori, alla violenza sessuale, alla violenza sessuale sui minori,

sentenza della Corte costituzionale, che ha definito che in questi casi l'alternativa alla custodia cautelare in carcere debba essere mantenuta. Ricordo un'altra misura importante, di cui abbiamo già parlato a suo tempo, quando abbiamo approvato questo provvedimento. Mi riferisco all'adozione della misura del braccialetto elettronico, prevedendo addirittura che il giudice debba specificare perché, in caso di custodia cautelare, non si sia preferita la misura delle procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1, cioè appunto la misura del braccialetto elettronico.

custodia cautelare ma, anche a fronte dell'esistenza di situazioni davvero di lieve entità di trasgressione dell'obbligo di dimora

la revoca di quella misura. Termino con un riferimento alla seconda parte del titolo di questo disegno di legge, che mi sembra una misura molto importante, cioè l'estensione della possibilità

lavorare di più sul tema delle relazioni famigliari, sul tema dell'accesso dei famigliari in carcere, sul tema delle telefonate dei detenuti alle proprie famiglie, sul tema della possibilità che la permanenza in carcere possa rappresentare non un momento di lacerazione degli affetti famigliari famigliari e delle relazioni sociali. Deve essere un momento in cui, all'interno del processo rieducativo, la famiglia, la relazione sociale, il gruppo di riferimento possano diventare un elemento della rieducazione e del reinserimento sociale delle persone recluse.

ma anche della sospensione della esecuzione della condanna. Come diceva giustamente il senatore Barani, la questione è stata dibattuta lungamente ed il Senato aveva introdotto anche la disposizione poi eliminata dalla Camera. C'è però da dire - come il relatore si è permesso sempre di osservare - che le valutazioni prognostiche sono sempre dei paletti estremamente inefficaci all'emissione dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere, soprattutto allorquando la valutazione prognostica debba abbracciare fatti che si verificano dopo la condanna. L'articolo 656 del codice di procedura penale è, per l'appunto, una norma dedicata alla esecuzione, la norma di apertura

quasi impossibile rimproverare a chiunque e, per altro verso, si tratta di vicende che, rispetto alla fase iniziale del processo, si caratterizzano per l'intervento di fatti obiettivamente del tutto imprevedibili. Quindi, si tratta, per un verso, di una norma che non avrebbe certamente funzionato e, per altro verso, di una richiesta di giudizio prognostico certamente impossibile. Passo al tema delle presunzioni, ossia al terzo comma dell'articolo 275. Vi sono tanti emendamenti al riguardo o, meglio, un maggior numero rispetto ai pochi emendamenti presentati. c'è da chiarire un aspetto. Il senatore Lo Giudice è appena intervenuto sull'argomento. Mi permetto di dedicare alla questione soltanto poche parole. Il fatto che, per un reato, non si preveda l'emissione obbligatoria della custodia cautelare in carcere certo non significa che detta misura non possa essere disposta. disposta. Si passa da un regime di obbligatorietà ad un regime di facoltatività. Il giudice è lasciato libero di valutare se per quel fatto, per come si è realizzato per quella personalità e per come essa si manifesta attraverso l'esame delle modalità di esecuzione del fatto, dei suoi precedenti eventualmente specifici, sia necessario intervenire con un provvedimento così drastico. Aver escluso, dal terzo comma dell'articolo 275 determinati reati non significa che, per quegli stessi reati, non possa essere instaurata la custodia cautelare in carcere. C'è poi da osservare - e qui do una risposta, permettendomi di non darla nel corso delle dichiarazioni di voto in sede di votazione dei singoli emendamenti - che questa materia è in maniera assolutamente completa da numerose sentenze della Corte costituzionale, la penultima delle quali è la sentenza n. 57 del 2013

Con questa ultima sentenza, sostanzialmente si chiude una stagione della Corte costituzionale che si è reiteratamente pronunciata, escludendo

Pertanto, è impensabile che il Parlamento possa reintrodurre disposizioni che la Corte costituzionale ha escluso dal novero dei reati inclusi all'interno del terzo comma per esempio - al concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte costituzionale ha ripreso una nota giurisprudenza della Corte di Cassazione, affermando che il concorrente esterno interviene occasionalmente, laddove la presunzione deve lambire contesti associativi caratterizzati da partecipazioni permanenti. Proprio nello spazio caratterizzato dalla differenza concettuale tra partecipazione permanente (chi partecipa quotidianamente) e vicende occasionali si trova anche la risposta all'impossibilità di introdurre il 416-*ter*, il cosiddetto voto di scambio, che è caratterizzato, per l'appunto, da partecipazioni occasionali legate a vicende di natura elettorale.

per il collegio di disporre un differimento di ufficio per vicende particolarmente complesse. A noi era sembrato che tale disposizione fosse ragionevole, quindi non

disporre anche un termine maggiore per la redazione della motivazione e il suo successivo deposito. La Camera ha ritenuto che il tribunale della libertà non potesse, d'ufficio, differire il termine della decisione né il successivo termine di deposito delle motivazioni a sostegno della decisione adottata; e lo ha fatto sulla base del principio che potremmo riassumere con il latinetto del *favor libertatis*. in terza lettura in Commissione, di non dover determinare un ulteriore ritardo nell'entrata in vigore di un testo che si stima evidentemente importante, necessario e tra l'altro simmetrico, se mi è consentito fare questo paragone, ai cosiddetti "svuota carceri". Noi dovevamo intervenire non soltanto sulle condanne, ma anche sulle custodie cautelari perché le statistiche del Ministero della giustizia, che per noi sono un punto di riferimento ovvio, davano indicazioni in ordine ad un numero eccessivo di detenuti in fase di custodia cautelare. Quindi tale norma si inserisce in un'iniziativa legislativa intrapresa da questo Parlamento potremmo dire al suo esordio, allorquando

ossia un numero eccessivo di detenuti. D'altronde i risultati sono arrivati se è vero, com'è certamente vero, che vi è stata una riduzione di 11.000

della legge introduttiva della tipicizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati, relativa al caso di un magistrato, o per meglio dire di un collegio, che avesse depositato un provvedimento *de libertate* in tempi successivi a quelli perentori entro i quali il provvedimento deve essere depositato, determinando la perdita di efficacia del provvedimento

per tale superamento di termini perentori fosse, per come effettivamente è, la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare e che pertanto già vi fosse una sanzione per il caso del ritardo, sanzione dotata, credo io, di una maggiore pregnanza rispetto alla previsione di un illecito disciplinare che, ripeto concludendo, esiste già nella lettera

condanna definitiva, è un tema certamente complesso e si riflette molto nei dati che ha fornito il senatore Lo Giudice che che evidenziano che nelle nostre carceri vi è una percentuale particolarmente alta di detenuti in custodia cautelare. Questo provvedimento punta proprio ad offrire una risposta a tale problema, ma va visto

tocca un punto che secondo me sarà fondamentale affrontare, che è quello della prognosi. È infatti evidente che si delega al giudice un'analisi prognostica in ordine

che recita: «Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi». Attraverso questa indagine si andrà a valutare il percorso che ha toccato le varie misure cautelari. infine alcune considerazioni svolte dal senatore Barani, per dire che è vero che il nostro ordinamento prevede un rimedio, l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione,

un passo avanti del Parlamento e delle Commissione parlamentari che lo hanno istruito con molta attenzione. Soprattutto, lo ripeto ancora una volta, si tratta di un provvedimento che va visto in combinazione con il decreto-legge n.

All'articolo 4 sono previsti i casi di custodia cautelare automatica, ovvero casi in cui ricorrono reati gravi per i quali si ritiene applicarsi la custodia cautelare «salvo

Inoltre, proprio per il tipo di altissima pericolosità di alcune fattispecie criminose, con l'emendamento successivo 4.101 noi proponiamo d'introdurre tra i reati per i quali si può applicare automaticamente la custodia cautelare della Repubblica n. 309 del 1990 (ovvero la legge sugli stupefacenti). L'articolo 74 prevede ipotesi di reato relative all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Signor Presidente, l'articolo 5 di questo provvedimento, così come era stato approvato dal Senato della Repubblica, prevedeva un'eccezione, nell'applicazione di quanto previsto in questa modifica del regime della custodia cautelare,

Mi chiedo, e vi chiedo, come mai ogni qual volta il Parlamento si trova a legiferare su questo articolo del codice penale, il 416-*ter*, le modifiche vengono sempre poste al ribasso. al ribasso. Naturalmente, al ribasso della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dei responsabili di questo che è uno dei peggiori reati previsti nel codice penale, ossia lo scambio elettorale politico-mafioso: io vengo eletto grazie ai voti richiesti alla mafia.

a quest'articolo, così come per altri che vengono citati (l'articolo 270 sul terrorismo e i reati connessi, e anche l'associazione mafiosa), per l'applicazione di questo regime che, naturalmente, si voleva limitare in presenza di casi di reato così gravi come questo. La portata dell'emendamento 4.2, che sto illustrando, tende semplicemente a reintrodurre questa

anche con l'espressione di preferenze. Saranno dunque migliaia i candidati che, nelle sette Regioni italiane, si confronteranno ancora una volta con un voto espresso con le preferenze. Quale migliore occasione

le misure cautelari personali debbano essere applicate con la misura custodiale più severa, ovvero quella del carcere? Perché non riparare al danno fatto dalla Camera nella parte in cui ha escluso l'articolo 416-*ter* da queste categorie di reati? L'emendamento 4.4 mira quindi a sanare il *vulnus* inferto dalla Camera a questo provvedimento di legge, facendo sì che lo scambio elettorale politico-mafioso

di congruità della detenzione carceraria in luogo di quella domiciliare. L'emendamento 4.3 mira invece ad inserire nella medesima categoria di reati anche quelli contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. Per questo tipo di reati noi chiediamo che valga la presunzione che ammette la prova contraria - per cui la misura della custodia cautelare sia quella carceraria e non domiciliare. Questo non perché siamo dei pazzi giustizialisti che vogliono le carceri piene, anzi: ricordo

entro il quale il tribunale deve prendere una decisione motivata, evitando così le due alternative che restano, cioè prendere una decisione affrettata senza aver letto le carte (quando naturalmente il caso sia particolarmente complicato) o lasciare decorrere i termini con conseguente cessazione degli effetti della richiesta di custodia cautelare, che magari in qualche caso, proprio perché il caso è complesso, sarebbe opportuno che rimanesse.

non praticare le procedure adeguate previste dal codice di procedura penale nei tempi previsti, determinando perciò la scarcerazione di persone perché non è stata trasmessa la documentazione. Sarebbe normale che ciò costituisse un illecito disciplinare. Qualunque professionista o funzionario che lasciasse decadere un termine importante, che determina addirittura la nullità di una atto che si presume motivato (perché altrimenti non sarebbe stato neppure richiesto), sarebbe sicuramente, come minimo, sanzionato disciplinarmente. Sarebbe quindi logico che lo fosse anche il magistrato inadempiente;

Forse questo sembra un po' appannato, ma noi riteniamo che anche questo provvedimento possa rientrare in quella deleteria politica di gestione della situazione carceraria, con tutta la serie dei vari svuota carceri.

custodia cautelare. Quest'ultimo è sicuramente un istituto utile e importante, che dà un grandissimo segnale non solo nei confronti dei criminali, ma di certo anche nei confronti delle persone offese dal reato, che almeno possono vedere prendere una posizione immediata da parte della giustizia. Se poi teniamo conto dei tempi e delle lungaggini processuali, probabilmente la migliore soddisfazione che può avere la persona offesa è proprio quella di vedere applicata subito la custodia cautelare. Ciò invece non accade o non accade bene. Infatti, fino a qualche tempo fa la popolazione carceraria contava una percentuale molto elevata di detenuti in custodia cautelare. Questo probabilmente per un abuso dell'istituto. Ebbene, noi non vogliamo assolutamente che vi siano forme di anticipazione della condanna; forme in cui l'espiazione della pena possa avvenire in un momento così precedente e magari a volte anche ingiusto.

Sotto questo profilo condividiamo le perplessità in ordine all'applicazione di questo istituto, ma non per la mancanza di bontà dell'istituto in sé, quanto per le problematiche connesse all'interpretazione delle norme e quindi all'applicazione dell'istituto nel concreto. Noi riteniamo, come abbiamo sempre ritenuto e sostenuto, che occorra sì una riforma della carcerazione preventiva, ma non che si arrivi al punto di valutare uno smantellamento dell'istituto della custodia cautelare. Non è il momento di parlare di smantellamento del rigore delle norme penali e delle norme di procedura penale.

Arriviamo a questo disegno di legge quando già le carceri sono state parzialmente svuotate, e questo grazie ad un insieme di provvedimenti che noi abbiamo fortemente osteggiato; osteggiato; quei provvedimenti che hanno portato alla liberazione anticipata, all'applicazione degli arresti domiciliari e alla previsione istituzionalizzata della reclusione domiciliare come una delle pene.

deleteri sono stati adottati da questo Governo e dalla sua maggioranza non per ristrutturare e riformare il sistema del diritto penale e della procedura penale, ma con il solo e unico obiettivo di risolvere un problema, tra l'altro tra l'altro emergenziale, relativo al sovraffollamento carcerario; problema che poteva essere affrontato in ben altra maniera, magari anche sfruttando progetti che erano già nati e che esistono già da anni,

di becera xenofobia, mentre alla fine si capisce che sono provvedimenti utili da farsi. Quando lo dice la Lega, però, sembra sempre una cosa brutta e sporca, mentre quando viene fatta dagli altri è la cosa più ragionevole del mondo.

ma che alla fine nasconde ipotesi certo non da poco. Purtroppo, abbiamo visto bocciare due nostri emendamenti che ritenevamo molto importanti. È vero che la custodia cautelare dev'essere applicata in presenza di alcuni requisiti e infatti, se si parla di questo, devono esserci esigenze cautelari: a nostro avviso, una delle migliori esigenze cautelari è dare risposta

intervento ci ha comunicato dei dati ancora più drammatici, dicendo che negli ultimi decenni lo Stato ha pagato 580 milioni

con capacità e scrivendo nell'articolo 27 della Costituzione che le pene non possono consentire trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, cosa che invece non avviene.

Poi, cari colleghi, c'è la legge Pinto, che viene applicata a qualsiasi organo in azione disciplinare, e cioè chiunque crei un danno allo Stato, lo Stato paga e poi c'è l'azione disciplinare nei confronti di chi ha sbagliato. Perché questo non viene applicato ai giudici? Perché la legge Pinto, cari colleghi, non viene applicata anche alla giustizia? Perché, signor Vice Ministro, non accade questo? Significa rispettare la Costituzione? Siamo tutti uguali di fronte alla legge oppure no? No, non siamo uguali,

nei confronti di chi ha sbagliato ed ha messo in carcere 23.000 persone, come ci ha detto il vice Ministro, che abbiamo risarcito con quasi 600 milioni di euro,

lampante. Ma perché non la applichiamo anche ai magistrati, che portano a morte in carcere, che è la morte giudiziaria, migliaia di persone ogni anno ingiustamente detenute? Ha ragione Pannella quando fa lo sciopero della sete e della

a capire quella che è la filosofia della nostra Costituzione, che ovviamente ci porta a dire che dovevamo avere più coraggio e non dovevamo prendere lezioni dalla maestrina della Camera, perché se la media dell'Unione europea, caro senatore Lo Giudice, è del 21,5 per cento di custodia cautelare in attesa di giudizio, noi non possiamo avere il 34,8 per cento, perché significa che in Italia non funziona. Non possiamo avere un sovraffollamento carcerario alla Auschwitz

un po' è meglio di niente e un bicchiere d'acqua è meglio che morire di sete, il nostro di oggi è un no politico perché non possiamo prendere lezioni da chi non ha né la cultura, né la capacità, né soprattutto la storia,

Presidente, intervengo brevemente, anche perché buona parte delle considerazioni politiche su questo testo le abbiamo già fatte in seconda lettura e perché le modifiche che sono state apportate dalla Camera a nostro avviso non snaturano il testo e quindi

Naturalmente molte considerazioni sono state già fatte in passato, in particolare sul numero molto alto di detenuti sottomessi a regime di custodia cautelare nel nostro Paese, anche in attesa di primo giudizio, e su

che dal nostro punto di vista sembra condivisibile su questo provvedimento. Questo provvedimento è un'inversione di tendenza rispetto a un andazzo che da molti mesi a questa parte attraversa il Parlamento del nostro Paese. Paese. Secondo questo andazzo l'unico modo per risolvere i problemi del Paese è aumentare le pene e farlo in maniera anche molto considerevole e pensare sostanzialmente che l'unica risposta ai problemi dell'Italia è il carcere.

ma il punto di fondo che noi vorremmo sottolineare è quello che invece a noi, nonostante tutto, il dettato costituzionale ci sembra ancora molto avanzato. avanzato. I Padri costituenti quando immaginarono il carcere come estrema *ratio* non erano diventati buonisti. Evidentemente, l'avevano fatto perché avevano colto alcuni aspetti di fondo della società di questo Paese e avevano studiato le legislazioni del mondo più adeguate. Erano figli di una stagione politica molto particolare e avevano compreso che le grandi questioni aperte nel nostro tempo non si risolvono semplicemente attraverso la repressione,

comminazione di pene spesso molto severe, soprattutto per i socialmente meno garantiti, sia essa stessa un tema di risoluzione dei problemi del Paese ci sembra una profonda degenerazione culturale. A noi piacerebbe discutere di questo con il Ministro e anche

siano solo gli anni di carcere che vengono commisurati? È possibile che lo Stato democratico rinuncia aprioristicamente a immaginare se possono esistere altre soluzioni capaci di produrre risultati migliori nel contrasto alle forme di criminalità organizzate e non? Questa è la domanda di fondo che noi ci sentiamo di porre. Sappiamo bene che è una domanda complessa,

Negli anni passati, quando gli Stati erano un po' meno democratici, utilizzavano il famoso adagio «Feste, farina e forche». Noi non vorremo che, siccome in questa fase storica storica c'è la crisi economica e, quindi, di soldi per fare le feste non ce ne sono e non c'è nemmeno troppa farina da distribuire, si usi solo la forca come elemento e strumento di calmieramento sociale per gettare in pasto all'opinione pubblica qualche elemento di propaganda. Faremo una battaglia culturale da questo punto di vista. La cominciamo oggi; l'abbiamo cominciata in questi mesi votando a favore di questi provvedimenti. Insisteremo sul tema che le questioni aperte nel nostro Paese, anche quelle così delicate di cui discutiamo stamattina, non si risolvono semplicemente con le strette repressive, le quali hanno un'utilità ovviamente, ma devono essere contestualizzate in una dimensione più ampia, cui, invece, il nostro Parlamento nazionale ha completamente rinunciato a discutere da molti anni a questa parte. Se oggi la giustizia italiana appare agli occhi dei cittadini come una cosa lontana, separata e un magma indistinto dentro il quale il più debole rischia di essere in difficoltà e il più forte rischia di cavarsela è anche perché il Parlamento ha rinunciato del tutto in questi anni a svolgere questa riflessione che, a nostro avviso, è serissima.

John Adams, secondo Presidente degli Stati Uniti (da non confondere con John Quincy Adams, sesto Presidente degli Stati Uniti), nel dicembre 1770, difendendo dei soldati britannici dopo il massacro di Boston, usò un'espressione «*Facts are stubborn things*», i fatti sono argomenti testardi. i fatti drammatici che riguardano il nostro caso sono questi: nel febbraio 2015 erano detenuti nelle carceri italiane circa 54.000 cittadini. Tra questi, quasi la metà, il 42 per cento (oltre 23.000 persone), sono detenute per ragioni cautelari, vale a dire senza una condanna che giustifichi la loro privazione della libertà. nei Paesi con cui abbiamo rapporti di vicinato ha una percentuale superiore alla nostra, il 60

Quasi la metà dei nostri concittadini sono quindi detenuti per ragioni cautelari. signor Ministro, sia uno Stato di Polizia, non uno Stato di diritto o di giustizia. prevede che ciascuno di noi, anche se sottoposto ad indagini o sia in corso un processo a suo carico, sia ritenuto innocente fino a sentenza passata in giudicato. Quella che ho descritto è la drammatica situazione a cui questo provvedimento tende, con lacune, con limiti, ma certo con buone intenzioni, a porre rimedio. E come lo fa?

si deve considerare l'aspetto della cautela nei riguardi di un pericolo, di quello che può avvenire se queste misure alternative non venissero adottate. Diverso è il caso di un evento di danno. Oltre agli indizi di grave colpevolezza, che esistevano anche prima, oltre all'aspetto dell'inquinamento probatorio, che riguardava la concreta possibilità che potesse avvenire, si è introdotto un altro aggettivo che ha un rilievo fondamentale nell'apprezzamento della validità delle motivazioni ed è che l'inquinamento probatorio sia considerato un fatto di attualità. Abbiamo avuto in molti casi alcune motivazioni per interventi privativi della libertà personale per fatti risalenti ad anni precedenti. Difficile immaginare un inquinamento probatorio per fatti su cui si indagava, risalenti a quattro o cinque anni precedenti; il pericolo di fuga, la reiterazione del reato e per ipotesi accusatorie che abbiano come previsione di pena una sanzione non inferiore ai cinque anni.

quando altre misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari, il braccialetto elettronico o altri fatti di questa natura, possono sopperire alle esigenze di cautela, di uscire da una situazione di pericolo, come si diceva prima, senza intervenire sulla privazione della libertà. è rafforzata la dimensione della motivazione per l'adozione di provvedimenti così afflittivi, e non solo della motivazione del pubblico ministero ma della autonoma motivazione del giudice che decide sulla richiesta del pubblico ministero per l'applicazione di misure cautelari; cosa che non è quasi mai avvenuta. Il giudice per le indagini preliminari, per la maggior parte dei casi, non ha fatto altro che sottoscrivere, senza alcun accertamento dei fatti, le ipotesi motivazionali del pubblico ministero.

nel caso dell'impugnazione, per cui è previsto un termine perentorio, non più ordinatorio cioè privo di sanzioni. In questo caso la sanzione prevista è l'inefficacia del provvedimento di sottrazione della libertà.

ove venisse riscontrata, com'è accaduto in 25 anni per 23.000 casi con quasi 600 milioni di indennizzo da parte dello Stato, l'obbligatorietà della attivazione dell'azione disciplinare nei riguardi dei giudici che si fossero resi responsabili di fatti gravi quali la privazione arbitraria e ingiusta della libertà dei nostri concittadini.

il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento ma vorrebbe anche, e mi faccio interprete di tale esigenza nei brevi secondi che mi separano dalla conclusione, il provvedimento che è stato cassato dalla Camera e che permette al "giardiniere" - cioè al Ministro della giustizia - di tosare la siepe quand'è in rigoglio eccessivo, e cioè che nel caso di un'azione strabordante della magistratura, a volte abusiva come nei casi che ho descritto, faccia sino in fondo la sua parte perché questo non avvenga e si contenga in uno Stato di diritto quello che i fatti testardi hanno dimostrato essere diventato il numero di cittadini privati della libertà senza cause legittime perché questo avvenga) uno Stato di polizia. Signor Presidente, nel primo passaggio parlamentare il Movimento 5 Stelle aveva votato a favore di questo disegno di legge. Adesso siamo chiamati ad un secondo voto sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, modifiche che, a nostro modo di vedere, sono peggiorative soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei reati per i quali vale la presunzione di adeguatezza della misura cautelare personale carceraria. L'abbiamo già detto prima ed è il caso di reiterare questo messaggio e questa motivazione. Tra poco più di un mese migliaia di candidati in sette Regioni italiane e altrettanti, e forse ancora più, in centinaia di Comuni, andranno al voto.

dal novero dei reati per i quali vale la presunzione di adeguatezza della misura carceraria invece di quella domiciliare in sede cautelare, è un grande punto interrogativo,

organizzata di tipo mafioso. Pensiamo che tutto questo sia incomprensibile per la stragrande parte dei nostri concittadini, è una decisione che va fortemente stigmatizzata ed è il motivo per il quale il Movimento 5 Stelle non voterà favorevolmente al provvedimento, per non dire del mancato accoglimento di un nostro emendamento, che avrebbe previsto anche i reati contro la pubblica amministrazione nel novero dei reati per i quali comminare la pena carceraria, in caso di sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per per irrogare una limitazione della libertà personale prima di un giudizio. Anche per i reati contro la pubblica amministrazione il Senato ha detto no. Se il Senato dice di no a queste misure, virtuose e necessarie per la pulizia di questo Paese, se i partiti, nonostante il chiacchiericcio, i «blabla» e i proclami, ancora non si decidono ad intraprendere la strada coraggiosa di una vera pulizia interna una vera selezione meritocratica e slegata dagli interessi più torbidi, questo Paese non cambierà. Noi continueremo, con il nostro impegno coerente, a voler offrire soluzioni, che talvolta sono state accolte, come talvolta noi abbiamo accolto proposte provenienti dalla maggioranza ma in questo caso veramente non possiamo votare favorevolmente.

detenuti in carcere in attesa di giudizio. Di questi molti (s'intende dire migliaia) saranno dichiarati innocenti dalla giustizia

Il carcere inadeguato, per quanto possa magari soddisfare qualche pulsione forcaiola, fa sì che dominino i delinquenti peggiori. Le persone che potrebbero magari davvero redimersi (perché questo dovrebbe essere lo scopo del carcere) o che non hanno nulla di cui redimersi

dei peggiori criminali detenuti in carcere, magari proprio di quelli che appartengono a qualche forma di delinquenza organizzata. Per porre rimedio a questa situazione, che pone l'Italia al secondo peggior posto come è stato già detto, tra i Paesi che dovrebbero essere più evoluti specialmente dal punto di vista della

Parlamento, e voteremo a favore anche oggi, pur sapendo che si sarebbe potuto fare di meglio e pur sapendo che il vero problema è la durata dei processi. La durata dei processi è fonte di un grave peso dal punto di vista anche finanziario. Conosciamo i dati diffusi poche settimane fa dal Ministero della giustizia sui 580 milioni già pagati di risarcimento per i processi troppo lunghi e per la detenzione ingiusta. Altri

il fatto che contemporaneamente si stiano approvando diverse misure che portano a un allungamento spropositato prescrizione, indegno di un Paese civile, fa sì che si ottenga esattamente l'effetto opposto. Avremo processi più lunghi perché il magistrato, giustamente, quando deve

Quanti casi, sia quelli testimoniati dalle statistiche, che lo stesso Ministero della giustizia fornisce, sia quelli testimoniati dall'esperienza delle cronache si risolvono con un'assoluzione? Il processo serve proprio a questo.

nella direzione giusta. Ci sono delle buone intenzioni e delle riformulazioni di determinati articoli che dovrebbero garantire maggiormente contro l'abuso della

concreto viene considerato grave e così sarà per le varie aggettivazioni introdotte oggi. Purtroppo sono state espunte alcune misure di grande buonsenso, oltre che di grande giustizia.

non si capisce bene perché. In un momento in cui bisogna raddoppiare, quadruplicare e decuplicare le pene per tutti ed allungare di decenni quella pena accessoria ed ingiusta che è un processo troppo lungo,

a favore dei magistrati che fanno il loro dovere e contro coloro che invece lasciano colpevolmente scadere dei dei termini, con la conseguente liberazione di persone che il magistrato stesso ha chiesto che fossero custodite in carcere, per cui si presume che ci fosse un buon motivo per farlo. Aggiungo un particolare importante a proposito di altri provvedimenti. Il Governo ha lasciato scadere la delega per l'attuazione di una norma approvata in passato che configurava la custodia domiciliare come forma principale - naturalmente non esclusiva Il Governo così veloce, così rapido e scattante ha lasciato scadere questa delega. Peccato.

Cesare Beccaria scrisse pagine straordinarie di cui dovremmo davvero ricordarci ogni giorno. In particolare, scrive che la pena, la detenzione prima del processo deve essere circoscritta

ci siamo dimenticati: non se ne dimenticano i 20.000 detenuti che sono in carcere senza mai essere stati condannati.

ci apprestiamo a votare questo disegno di legge, che la Camera ha varato ed il Senato ha corretto. Ci troviamo ora in terza lettura, cercando di dare un'ulteriore risposta alla sfida delle sfide: fare in modo risposta alla sfida delle sfide: fare in modo che il nostro sistema carcerario sia in grado di rispondere

alla dimensione delle garanzie e alla dimensione della sicurezza. In un Paese moderno, avanzato, civile, a democrazia matura, sicurezza e garanzie devono procedere insieme: squilibrare queste due dimensioni non va bene. L'Italia, l'italietta, ha saputo fare anche questo. In questi mesi, grazie all'azione del Governo e della maggioranza, grazie anche ad un dialogo serrato e forte con l'opposizione, abbiamo cercato di dare una risposta al sovraffollamento carcerario in grado di tenere insieme garanzia e sicurezza.

sottoposto a procedure di infrazione da parte dell'Europa, sottoposto alla derisione e ad un giudizio severo sia nel campo dei diritti umani che in quello della tutela della sicurezza, ad esempio con l'aggiramento continuo del 41-*bis* da parte delle organizzazioni mafiose. Colleghi, ricordo a tutti che partivamo da una situazione veramente preoccupante e drammatica. A marzo 2013, il totale dei detenuti presenti nel nostro sistema carcerario era pari a 65.831 detenuti.

Per la prima volta non si è imboccata questa strada e si sono ottenuti risultati permanenti e duraturi. Questo risultato non ha messo in pericolo la sicurezza del Paese Paese e non ha creato quello che molti paventavano stracciandosi le vesti e gridando «al lupo!», cioè che il nostro Paese sarebbe stato invaso da un aumento dell'indice di criminalità. è stato fatto con un lavoro misurato e progettuale, in grado finalmente di tenere insieme - come dicevo all'inizio - sicurezza e garanzie. anche un altro problema nell'ambito del sovraffollamento, quello della custodia cautelare. Il nostro Paese spicca anche per questo dato negativo: la custodia cautelare non era l'eccezione, ma via via nell'italietta stava diventando la regola.

Ma 18.696 è ancora un numero elevato; ecco allora l'intervento di oggi, che ci apprestiamo ad approvare. La custodia cautelare non diventa più la prima misura, ma diventa una misura rigorosa e misurata realmente da un lato con la gravità dei reati e, dall'altro, con una condizione necessaria e indispensabile di cui il nostro sistema di sicurezza non può fare a meno. Non diventa quindi una misura

quindi non un pericolo generico che cammina con il tipo di reato. Abbiamo voluto prevedere che anche per il pericolo di fuga, come per la reiterazione del reato debba esserci un'attualità concreta e debbano essere motivati. In questo senso, la scelta che il relatore ha spiegato in diversi interventi qualifica e mette insieme sia la domanda di garanzie sia la richiesta di sicurezza ed evita il bisticcio tra queste due fondamentali condizioni di una democrazia avanzata. Cari colleghi, penso che questa sia una scelta indovinata e qualificante. Ce n'è stata un'altra che è stata valutata bene ed è fondamentale: quali sono i reati per cui è necessario attuare l'obbligatorietà della custodia cautelare? Normalmente sono quelli che via via stiamo provando a descrivere sotto la lezione storica che Falcone ci ha consegnato, che è quella del doppio binario: i reati di sovversione, di terrorismo e quelli di mafia. Per questi tipi di reati la domanda di sicurezza è forte e qualificante e quindi c'è obbligatorietà della custodia cautelare. Per gli altri reati, alcuni dei quali

e quindi di mettersi in condizione di rispettare e mettere in equilibrio sicurezza e garanzia. Quindi, anche in questo caso nessuna via di fuga per chi pensa di poter utilizzare alcuni tipi di reati per non incorrere nel rigore della legge.

Abbiamo scelto la via della depenalizzazione: una via moderna e avanzata che il nostro Paese aspettava da venti, trent'anni; la via della messa alla prova, la via di ammodernare il nostro sistema carcerario. Dobbiamo continuare su questa strada senza ledere un Paese, diritto di nuova generazione e diritto moderno e avanzato che è quello della sicurezza. È una strada che dobbiamo continuare

La 14ª Commissione, in connessione con l'indagine conoscitiva deliberata il 18 settembre 2013 sul tema della proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo, ha svolto in sede informale numerose audizioni di approfondimento con gli ambasciatori accreditati presso la Repubblica italiana di diversi Paesi (Egitto, Marocco, Giordania, Montenegro, Tunisia, Turchia e Malta), nonché con rappresentanti di enti di ricerca (IAI, ISPI, CESPI e CESI), con il Presidente della Camera commercio italo-araba ed i direttori per l'integrazione europea e per i Paesi del Mediterraneo e del Medioriente del Ministero degli affari esteri.

prende le mosse dalla sentita esigenza di rifocalizzare l'attenzione politica delle Istituzioni dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri sulle problematiche del Mediterraneo, inteso come quadrante strategico per la stabilità politica ed economico-commerciale europea e mondiale. della giusta e necessaria enfasi posta sugli ultimi allargamenti dell'Unione a Nord e a Est, nel 2004 e 2007, e del sostanziale esaurimento dell'iniziale spinta propulsiva del Processo di Barcellona, appare ora essenziale restituire centralità e priorità alla frontiera Sud dell'Unione, come auspicato anche dal Presidente del Consiglio nel suo intervento in Senato svolto in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015. considerando la rilevanza assoluta che riveste il Mediterraneo per l'Europa e per il mondo intero in termini di sicurezza, flussi migratori e rapporti economici e commerciali e considerata l'opportunità che una efficace politica euro-mediterranea puo` rappresentare per l'Unione europea quale attore globale sulla scena mondiale; necessario un profondo cambiamento nell'approccio dell'Unione europea nei confronti del Mediterraneo nel suo complesso che, come evidenziato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 3 luglio 2012, costituisce una macroregione che va considerata come un insieme coerente, un bacino unitario di riferimento, in cui sono condivise molte caratteristiche e priorità comuni, comuni, e che l'Unione europea debba elaborare nuovi paradigmi, nuovi approcci politici e nuovi strumenti d'azione, che pongano il tema del rilancio del Mediterraneo in termini diversi, più moderni ed inclusivi,

in *partnership* con i diversi livelli di governo, in modo da valorizzare le istanze sub-nazionali e le realtà associative, con la flessibilità necessaria a garantire la fattibilità dei programmi, oggi irrigiditi, nei modelli del Processo di Barcellona e dell'Unione per il Mediterraneo, dal livello statale e dai vincoli politici ad esso connessi, ponendo particolare attenzione ai progetti di cooperazione nel settore culturale e nei confronti delle nuove generazioni; Nei rapporti tra i Paesi dell'Unione europea e quelli della sponda meridionale ed orientale del Mediterraneo è necessario superare definitivamente la logica neocolonialista e fondare le relazioni su principi di parità e reciprocità, per consentire agli Stati membri della parte Nord del Mediterraneo di cooperare «paritariamente» con quelli della sponda Sud. Questi ultimi devono essere i veri protagonisti dei propri cambiamenti, necessari ad avanzare nella direzione della democratizzazione e dello sviluppo: a tal fine, occorre rafforzare la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, valorizzando i lavori dell'Assemblea parlamentare euromediterranea Altro aspetto fondamentale è la dimensione sociale e culturale del Mediterraneo, che costituisce un'opportunità concreta per la crescita economica ed il lavoro delle giovani generazioni, dove la cultura svolge un insostituibile ruolo di rafforzamento del processo di sviluppo e di valorizzazione degli aspetti di di comunanza e vicinanza tra i diversi popoli. A tal fine, occorrono azioni di intensificazione degli scambi culturali ad ogni livello della società civile e delle istituzioni, per esempio rafforzando il lavoro svolto dalla Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture, rafforzando i programmi di scambio tra studenti universitari, come Erasmus Mundus, creando occasioni di collaborazione nell'ambito della cultura, ad esempio attraverso produzioni teatrali, audiovisive e altro, e del patrimonio artistico e storico, istituendo programmi di collaborazione tra amministrazioni locali e regionali. Le due sponde del Mediterraneo presentano importanti aspetti di complementarità, dal punto di vista delle risorse materiali e immateriali di cui ciascuna è portatrice, che è opportuno valorizzare, per sviluppare le necessarie sinergie economico-produttive. A tal fine, può essere opportuno riprendere l'ipotesi della istituzione di una banca mediterranea, esplorando le diverse soluzioni adottabili, per promuovere investimenti diretti esteri nei Paesi del Maghreb e del Mashrek, sia al fine di sfruttarne le potenzialità di rendimento, sia al fine di ridurre il substrato di povertà e malessere, che contribuisce alla situazione di instabilità e al fenomeno dei flussi migratori. La profonda e prolungata instabilità nell'area del Mediterraneo ha, inoltre, reso ormai imprescindibile e urgente l'elaborazione di una reale politica comune europea in materia di flussi migratori che, in attuazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consenta all'Unione di agire in modo organico e integrato nei confronti del fenomeno dell'immigrazione illegale, non limitandosi ad affrontare i risvolti più emergenziali, ma aggredendo i meccanismi e le cause del fenomeno, integrando nella sua azione gli strumenti dell'Unione per il Mediterraneo, della politica di vicinato, del Servizio europeo per l'azione esterna, della cooperazione allo sviluppo, degli aiuti umanitari e gli altri strumenti economici e finanziari come il Fondo asilo, la ricostruzione e sviluppo (BERS). Cari colleghi, ai fini di un'efficace politica di gestione dei flussi migratori, sarebbe opportuno che gli accordi con i Paesi della sponda Sud, finalizzati al contrasto alle migrazioni irregolari e al rimpatrio dei clandestini, fossero negoziati e stipulati dall'Unione europea nel suo insieme, superando la logica degli accordi bilaterali. Al riguardo, si accoglie con favore l'intenzione espressa dalla nuova Commissione Juncker nel Programma di lavoro per il 2015 di sviluppare una nuova politica della migrazione e si auspica che in tale contesto sia attribuita la dovuta considerazione alle condizioni, particolarmente gravose, del fenomeno migratorio illegale, che interessa i confini marittimi meridionali dell'Europa, sia per gli stessi migranti clandestini, sia per le istituzioni e le comunità ove avviene il loro primo approdo, riconoscendo la specificità e la peculiarità di tali flussi migratori rispetto a quelli che interessano le altre zone dell'Unione europea. Sarebbe inoltre auspicabile anche un riassetto dell'attuale normativa in tema di protezione e asilo, al fine di migliorare le procedure e la redistribuzione degli oneri legati all'accoglienza, garantendo maggiore equità nell'impegno dei diversi Paesi dell'Unione e risposte più funzionali alle esigenze dei richiedenti. Peraltro, il 16 aprile 2014, si è svolta, ad Alicante, in Spagna, la prima riunione informale a livello dei Ministri degli affari esteri di Italia, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia, Malta e Francia del cosiddetto Gruppo Mediterraneo sul tema delle migrazioni irregolari. Si auspica che tale coordinamento tra i Paesi mediterranei dell'Unione europea possa utilmente rafforzare il coinvolgimento dell'intera Unione europea sul quadrante del Mediterraneo. È inoltre da considerare con favore la posizione assunta dal Consiglio Giustizia e affari interni, lo scorso 10 ottobre, sul tema «Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori», in cui si è delineato un approccio fondato su tre pilastri: la cooperazione con i Paesi terzi, con un'attenzione speciale alla lotta contro i passatori e i trafficanti di esseri umani; il rafforzamento della capacità dell'Agenzia Frontex di reagire con flessibilità e tempestività ai rischi e alle pressioni emergenti; le azioni dell'Unione europea atte a sostenere e dare piena attuazione al sistema europeo comune di asilo, anche attraverso una maggiore cooperazione operativa. Sarebbe inoltre utile approfondire l'ipotesi di studiare la fattibilità di consentire - come già prefigurato dalla Comunicazione della Commissione europea «Una *task force* per il Mediterraneo» che le domande di asilo possano essere presentate presso una delle rappresentanze diplomatiche dell'Unione ubicate nei Paesi terzi di partenza o di transito dei flussi, evitando così, ad esempio, le drammatiche traversate del Mediterraneo e recidendo l'intermediazione della criminalità organizzata nella gestione di tali flussi. Da eventuali sviluppi in tal senso, conseguirebbe anche la possibilità di fronteggiare con maggiore severità l'utilizzo abusivo delle procedure

specifica della Tunisia, in cui la «rivoluzione dei gelsomini», che ha avviato i sommovimenti della «primavera araba», ha dato luogo a un processo di democratizzazione costituzionale, interna alla Libia, ove il vuoto istituzionale che ha fatto seguito al rovesciamento del regime precedente, ha dato spazio al riacuirsi delle contrapposizioni interne tra le principali fazioni di Tobruk, Tripoli, Misurata e Zintan, Qui si auspicherebbe davvero un intervento della Comunità europea come ruolo terzo per determinare l'assetto. Concludo con Concludo con una considerazione importante che la Commissione ha voluto svolgere per quanto riguarda il superamento del conflitto israelo-palestinese, che è un fatto di particolare importanza per la stabilità dell'area, e ricordando il recentissimo accordo raggiunto sulla questione del nucleare in Iran, che è un altro elemento di stabilizzazione che si è creato nell'area.

sugli avanzamenti ottenuti nella direzione di una rafforzata e rinnovata politica mediterranea dell'Unione europea e propone, a tal fine, l'istituzione di una sessione parlamentare annuale legata alle tematiche del Mediterraneo, a cui il Governo sarà chiamato ad intervenire.

un ringraziamento a lui e al senatore Martini, che hanno lavorato come relatori all'indagine conoscitiva sul Mediterraneo, ai membri della 14a Commissione, che hanno lavorato in termini di un confronto costruttivo e in un buon clima di approfondimento, e naturalmente alla Presidenza del Senato e ai Capigruppo,

d'accordo con le Commissioni del Senato e anche con quelle della Camera, su questo aspetto del Mediterraneo. Durante la Presidenza italiana di turno, ci siamo un po' suddivisi i compiti e il lavoro. È stato un lavoro

C'è un motivo, se volete formale, e c'è un motivo politico per cui abbiamo chiesto di fare questo confronto in Assemblea. Il motivo formale lo ha già spiegato il senatore Mauro. Avevamo presentato - e c'era stato anche un intervento del Governo

in modo specifico il ruolo del nostro Paese all'interno dell'Unione. È frequente tra noi un dibattito e una riflessione che hanno un fondamento. tema del ruolo e delle funzioni del Parlamento, oltre che nella riforma del bicameralismo, debba essere affrontato. Qual è il ruolo di un Parlamento moderno oggi nei confronti del Governo?

non stiamo facendo bene - questo è il mio giudizio - con continuità né l'uno e né l'altro. È un tema che dovremmo porci e saper affrontare. il Mediterraneo non può essere il grande tema su cui il Parlamento si impegna con continuità per poi periodicamente confrontarsi con il Governo, se vogliamo che l'azione del nostro Paese, che caratterizza un impegno politico del nostro Paese nell'Unione europea, abbia pieno successo e tutto il respiro necessario? Non è scontato. Vengo alla penultima considerazione. Se noi oggi

nello spazio del pranzo. Mi auguro che tutti non vadano a pranzo e che si partecipi a questa discussione. Questo ci dice come ci sia un serio aspetto di sottovalutazione del problema. In alcuni Stati europei il Mediterraneo viene visto come uno dei tanti mari che bagnano l'Europa. In altre situazioni si dice che il Mediterraneo si affronta quando la Presidenza di turno è di un Paese mediterraneo e poi quando invece non è del Mediterraneo si affrontano temi come l'Ucraina. Noi abbiamo voluto dare spazio nell'assemblea della COSAC all'Ucraina quanto al Mediterraneo, perché non c'è una suddivisione a seconda di chi esercita la Presidenza di turno. Il Mediterraneo - è l'ultima considerazione che faccio non è davvero uno dei tanti mari che bagnano l'Europa. Non è soltanto questo. Nelle rive Sud del Mediterraneo risiedono oltre 400 milioni di persone, molti giovani. Ci sono tensioni e speranze. Ci sono spiragli di pace e problemi irrisolti. Ci sono guerre, conflitti e azioni del terrorismo che non possono essere sottovalutate. Ci sono Paesi, come la Tunisia, che costruiscono una solida democrazia, e, comunque, su questo vanno aiutati dopo la primavera araba. Ci sono i processi in corso in Giordania. C'è il Marocco, che ha anticipato le primavere arabe costruendo una riforma costituzionale democratica significativa, ma c'è anche la Siria. C'è il conflitto che si è aperto nello Yemen e c'è la Libia. Ci sono infine gli annunci, che dobbiamo considerare positivi e sottolineare con forza,

non sono dei sinonimi, perché un'operazione di polizia internazionale può rendersi necessaria se lo decide la comunità internazionale, ma è mirata, *ad hoc*, non è un conflitto generalizzato e costruisce un dopo, tutela il rispetto dei diritti umani. ha senso quando si rende inevitabilmente necessaria, ha senso se è all'interno di un procedimento politico, di una strategia politica, di un'idea di politica e di diplomazia come quella prevalsa fino ad ora nelle trattative con l'Iran.

in relazione con il Governo, del problema del Mediterraneo in tutti i suoi aspetti - economici, ambientali, di conflitto, di stabilità, di costruzione della pace, di confronto e di formazione culturale e di ruolo stesso delle religioni - un tema che impegni

far vanto di se stessa, ma perché sono convinto sia la sua funzione nell'interesse dell'Unione europea. L'Unione europea, se vuole essere una democrazia sovranazionale, non può permettersi di sottovalutare o di delegare ad altri le responsabilità sul Mediterraneo. Deve assumersele tutte quante e in prima persona. Presidente, vorrei sottolineare ai colleghi un aspetto insito nelle parole pronunciate dal presidente Chiti

che i singoli Paesi procedano in ordine sparso a disegnare la loro politica verso il Mediterraneo; noi chiediamo che vi sia un approccio

chiediamo che il Parlamento italiano si faccia carico, anche nell'ambito dei rapporti interparlamentari che esistono, di una politica di buon vicinato tra l'Unione europea e gli altri mediterranei. Il presidente Chiti ha detto parole di verità e io non posso che sottoscriverle. In ogni incontro internazionale che noi ci troviamo a vivere

Il Mediterraneo è oggi tema centrale se l'Europa vuole avere un futuro, perché da esso vengono problemi ma possono venire opportunità. La politica europea non può delinearsi, su impulso in particolare dei Paesi del Nord - e della Germania, diciamo la verità, perché questa è la realtà - solo nello scenario del Nord Est europeo. Sappiamo che i problemi dell'Ucraina sono enormi: li abbiamo condivisi, abbiamo discusso profondamente in quest'Aula la situazione dell'Ucraina, della Georgia, dell'Azerbaijan e dell'Armenia. Sono questioni che viviamo giornalmente, ma il tema del Mediterraneo oggi è centrale. Consentitemi di

che vi è un cambiamento della politica e dell'approccio americano rispetto ai temi del Mediterraneo. Gli Stati Uniti d'America, in questi anni, si sono trasformati da Paese che aveva bisogno di approvvigionamento energetico in Paese esportatore. Pertanto l'Europa, oggi, deve assumere in prima persona la responsabilità della gestione di temi come quelli relativi al Mediterraneo e agli equilibri complessi che riguardano il Medioriente. Non c'è più, e ci sarà sempre meno, la tutela americana rispetto alle vecchie abitudini su cui ci siamo ripiegati. Ecco allora Ecco allora il punto: non è l'Italia da sola che può fare una politica di buon vicinato con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma è l'Italia che può chiedere all'Unione europea di farsi carico di una sensibilità nuova. Vi invito a fare una piccola ricerca negli archivi dell'Unione europea. In un anno abbiamo dato alla sola Polonia l'equivalente del complesso degli aiuti che sono stati dati in tutti questi anni all'insieme dei Paesi del Mediterraneo.

relazioni umane con i giovani universitari dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i Paesi rivieraschi dall'altra parte del Mediterraneo. Facciamo un grande Erasmus che colleghi questi giovani alle nostre università e che mandi anche i nostri giovani nelle loro università, che sono tempio di una cultura radicata e profonda. Non dimentichiamo, infatti, che nel Mediterraneo sono state capaci di misurarsi le grandi civiltà: dagli egizi, agli antichi greci, all'antica Roma, tutto è lievitato attorno al Mediterraneo che oggi, certamente, è anche mare di disperazione ma che noi dobbiamo riconvertire a mare di opportunità e collaborazione, di dialogo interreligioso, perché anche questa è questione

Il Governo è particolarmente grato per questa occasione, perché nelle ultime iniziative del ministro Gentiloni, ma già il nostro approccio è sempre stato quello di porre il Mediterraneo maggiormente al centro dell'iniziativa dell'Unione

in modo drammaticamente decisivo con la crisi in Libia e con quanto accaduto, anche di recente, in Tunisia, che ha ravvivato una attenzione da parte dell'Unione europea

Mi riferisco alla parte dove si dice che sarebbe opportuno, inoltre, approfondire l'ipotesi di studiare la fattibilità di consentire che le domande di asilo possano essere presentate presso una sede di rappresentanza diplomatica dell'Unione europea europea ubicata nei Paesi terzi di partenza o di transito dei flussi, evitando così - ad esempio - le drammatiche traversate del Mediterraneo e recidendo l'intermediazione della criminalità organizzata nella gestione di tali flussi. Da eventuali sviluppi in tal senso conseguirebbe anche la possibilità di fronteggiare con maggiore severità l'utilizzo abusivo delle procedure di asilo da parte di chi si trovi ad essere intercettato. Il documento del Consiglio n. 16045/13 ha affermato, infatti, che il 72,94 per cento dei migranti irregolari ha attivato le procedure per la protezione internazionale solo dopo l'intercettazione, circostanza che può essere valutata come un indicatore quantitativo di un abuso della procedura di asilo. In questo riconosciamo la presa di coscienza, che non possiamo che apprezzare, che quanto sta avvenendo oggi è molto differente rispetto alla semplice richiesta di asilo, che necessita invece di approfondimento serio in tempi rapidi. C'è un fronte di guerra innescato in tutta l'area mediorientale che si è esteso alla sponda Sud del Mediterraneo e che minaccia il nostro Paese da vicino. È altrettanto vero che il Mediterraneo non può essere semplicemente letto come una problematica legata ad aspetti economici. Si fa riferimento nel testo ad opportunità di promuovere investimenti diretti esteri nei Paesi del Maghreb. Questo è certo, ma giustamente - e come da tempo noi sosteniamo - l'aiuto deve arrivare innanzitutto laddove i problemi si generano, laddove l'economia mette le persone in difficoltà e dove poi si è aggiunta anche la questione della guerra. in queste ore il nostro Ministro degli esteri si è spinto a pensare anche ad un intervento militare, che rappresenta un salto di qualità in termini di coscienza e di partecipazione.

Troviamo nel documento dei giusti richiami al fatto che le politiche non possono essere limitate a scelte bilaterali: tra l'Italia ed altri Paesi piuttosto che tra alcuni Paesi europei ed altri Paesi del Mediterraneo. Troppe volte abbiamo visto sedersi ai tavoli di concertazione

che, come nella fase finale viene indicato, si invita il Governo a riferire almeno annualmente rispetto alla situazione della politica mediterranea e dell'Unione europea. Proporre una sessione specifica non è superfluo e non è un lusso. Abbiamo una situazione infuocata ai nostri confini. La gestione stessa dei flussi migratori non può essere ricondotta ai problemi dell'Italia, come se fosse un problema nazionale. Si tratta del confine europeo corretto che, all'interno della risoluzione, sia indicata la necessità che la politica europea nel suo insieme si faccia carico anche dei costi riguardo alla gestione dei flussi migratori. Approviamo quando, all'interno della relazione, si indica e si auspica che in tale contesto sia attribuita la dovuta considerazione alle condizioni particolarmente gravose del fenomeno migratorio illegale, che interessa i confini marittimi meridionali dell'Europa sia per gli stessi migranti clandestini sia per le istituzioni e le comunità ove avviene il loro primo approdo, riconoscendo la specifica peculiarità di tali flussi migratori rispetto a quelli che interessano altre zone dell'Unione europea. Sarebbe inoltre auspicabile anche il riassetto dell'attuale normativa in tema di protezione e di asilo, al fine di migliorare le procedure e la redistribuzione degli oneri legati all'accoglienza, garantendo maggiore equità nell'impegno dei diversi Paesi dell'Unione europea e risposte più funzionali alle esigenze dei richiedenti. Non sfugge in questo caso un salto di qualità in termini di coscienza. Il Governo deve prendere atto che, all'interno della Commissione politiche dell'Unione europea, queste riflessioni sono state svolte. Non è un problema che riguarda l'Italia, ma è un problema di cui tutta l'Europa deve essere investita. Se ci sarà questa presa di posizione, il nostro voto sarà decisamente favorevole. Ciò non toglie che non condividiamo quanto all'interno della risoluzione è indicato, in termini di favore, di consenso e di positiva considerazione, riguardo a Mare nostrum. Non condividiamo che nella risoluzione sia indicata la necessità di sostenere con forza l'iniziativa europea Operazione Tritone, che rappresenta il naturale sviluppo della positiva esperienza di Mare nostrum, attuata dal Governo italiano. Questa non è stata, e continua a non essere, una positiva esperienza. Continua a non esserlo per coloro che trovano la morte all'interno dei trasbordi fatti dalla criminalità, alla quale non possiamo prestare il fianco e alla quale, purtroppo, da troppo tempo il nostro Paese si è invece prestato, anche con una gestione che noi riteniamo scellerata dell'utilizzo delle navi militari nel trasportare immigrati clandestini da una parte all'altra del Mediterraneo, sostenendo quindi un'attività criminale.

nella parte in cui si chiede all'Unione europea di farsi carico della situazione e nella parte in cui si definiscono i tre pilastri: la cooperazione con i Paesi terzi, con un'attenzione speciale alla lotta contro i passatori e i trafficanti di esseri umani; il rafforzamento della capacità di FRONTEX di reagire con flessibilità e tempestività ai rischi e alle pressioni emergenti; le azioni dell'Unione europea atte a sostenere e dare piena attuazione al nostro sistema europeo comune di asilo, anche attraverso una maggiore cooperazione. Questo non è e non può essere un problema italiano. Da troppo tempo, invece, l'Italia è lasciata sola nella gestione di questo fenomeno,

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, signore e signori tutti, la risoluzione che viene sottoposta oggi all'attenzione di questa Assemblea prende le mosse dall'esigenza - condivisa in 14a Commissione - di riattualizzare l'azione politica delle istituzioni europee e dei suoi Stati membri sulle problematiche del Mediterraneo, anche nella prospettiva di un rafforzamento del ruolo strategico dell'Europa sullo scacchiere mondiale. È una frontiera, quella del Sud dell'Unione che, esaurito il pur giustificato allargamento degli orizzonti europei a Nord e ad Est, necessitato dalla caduta del muro di Berlino, soprattutto in questo momento storico, si propone con decisione per il suo rilievo strategico, ben oltre l'area che delimita. È dall'estrema labilità ed interdipendenza dei confini mondiali che discende per l'Europa una necessaria e diversa attenzione verso quest'area, e non solo per vedervi coinvolti temi in materia di sicurezza e di controllo dei flussi migratori o per privilegiare dei rapporti economici e commerciali, ma soprattutto per realizzare una politica europea più solidaristica nel Mediterraneo che, di fatto, rafforzerà la stessa Europa. Occorre però che l'Unione europea, da un lato, superi i modelli di certo bilateralismo interessato e, dall'altro, sviluppi nuovi modelli di cooperazione che valorizzino le comunità intra-nazionali e le diverse realtà associative, con una duttilità maggiore di quella iniziata nel 1995 con il Processo di Barcellona e proseguita nel 2008 con la costituzione dell'Unione per il Mediterraneo. In questa logica è decisivo, quindi, un approccio teso a riconoscere una comunanza sociale e culturale dell'area mediterranea, come imprescindibile strumento di rafforzamento di un diverso e più rispettoso processo di sviluppo dei rapporti tra i popoli, ed è altrettanto importante, nella nobiltà di tali intenti, evitare che si riproducano certi errori, interni oltre che esterni. Sarebbe profondamente sbagliato partire dal privilegiare certe visioni, tanto ideologiche quanto miopi, dell'economia di mercato, pensando che da esse e solo da esse - in modo non dissimile da certe ideologie esportatrici di democrazia occidentale tardo-imperiale - discendano automatici cambiamenti sociali, con relativo benessere accluso. Conosciamo bene il prezzo che si è pagato e che molti Paesi europei - compreso il nostro - stanno pagando per queste false certezze. Non basterà, quindi, solo pensare di creare una banca macroregionale, della quale si chiede

questa del Sud e del Nord dell'Africa, che il nostro Mezzogiorno conosce bene e che non ha mai trovato soluzione definitiva. La questione cosiddetta meridionale ha contribuito più a creare alibi nelle paternalistiche classi governative succedutesi nel tempo che conforto nelle popolazioni del Sud. Eppure questo popolo, il mio popolo, ha cercato, in questi lunghi lustri trascorsi dal dopoguerra risorgimentale, di affrancarsi dall'elemosina assistenzialistica e dalle false promesse, ma con alterne vicende, scandite anche dalle congiunture economiche e dalle crisi sociali, l'ultima delle quali, per alcuni versi peggiore di quella del '29, ci sta ancora piegando. Eppure questo popolo, il popolo del Sud Europa, è accomunato in un comune destino ai popoli che si affacciano sulla sponda opposta del Mediterraneo ed ha tutte le carte per poter osare: un grande bacino di manodopera, notevoli professionalità acquisite, risorse umane altamente qualificate. Sono tutte risorse caratterizzate dalla loro inutilizzazione. C'è ormai una classe di Governo nazionale ed europea che preferisce l'asservimento del Sud, di tutti i Sud, e un'altra locale che cerca di ricavare un utile personale da tale servitù. L'attuale Italia, provincia del Sud Europa, che condanna una zona così vasta del suo territorio, Sud del Sud, alla disperata marginalità nel perseguimento di politiche di pareggio di bilancio e di tassazioni inique, che impediscono ogni concreta iniziativa imprenditoriale, ha intenzione di cambiare questa prospettiva? Questa è anche la scommessa che si vuole vincere con la risoluzione in esame. Diversamente, come fare a credere ad un Paese, l'Italia (e quindi all'Europa), membro di una comunità di Stati che vuole farsi propugnatore dell'emancipazione di ciò che sta a Sud di se stessa e dell'Europa, quando non riesce ad emancipare il suo Sud? Eppure, proprio ora per affinità il nostro Sud, parte integrante del Sud del Mediterraneo, potrebbe costituire un ponte ideale e non un semplice approdo di disperati, una sorta di camera di compensazione tra le istanze dell'Europa continentale e quelle dell'area mediterranea. Potrebbe essere e diventare quell'opportunità di spostare il baricentro dell'Europa, decisiva per rilanciare le enormi potenzialità represse del nostro Mezzogiorno e quindi dell'intero Paese. Potrebbe essere l'inizio di un progetto per il nostro futuro come Europa, in cui far coesistere più centri d'azione e dove questa parte dell'Europa può cessare può cessare di essere ostaggio inerme di classi politiche parassitarie e gattopardesche e porsi in funzione di controbilanciamento di un'Europa germanocentrica. Una cosa certamente non si potrà più accettare: che il Sud possa essere messo al centro di guerre tra poveri, come è stato fatto con accordi bilaterali a livello europeo di pseudocooperazione agricola stipulati con Paesi mediterranei, dai quali hanno tratto beneficio, come al solito, solo i Paesi del Nord industrializzato. e solo in questa prospettiva, che trova ragione d'essere l'attuazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di cui tanti si dimenticano. Ecco allora che gli strumenti dell'Unione per il Mediterraneo, della politica di vicinato, del servizio europeo per l'azione esterna, della cooperazione allo sviluppo, degli aiuti umanitari e gli altri strumenti economici e finanziari come il Fondo asilo, migrazione e integrazione, la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dovranno andare oltre la frammentarietà degli interventi, dirigendosi con minore incertezza sul coinvolgimento complessivo dei Paesi del Sud del Mediterraneo, ma anche e soprattutto delle aree depresse del Sud Europa. Questi sono dei campi di investimento su cui speriamo si indirizzino le risorse richiamate dal piano Juncker. È in questo modo che si potrà realizzare il sostegno sincero ad un genuino processo di democratizzazione politica e sociale dei Paesi del Sud del Mediterraneo ed una loro definitiva affrancazione dal colonialismo. Permettetemi infine un'ultima annotazione, anche se non ve n'è traccia nella risoluzione. Mi riferisco alla mancata soluzione dello storico conflitto israelo‑palestinese, che è ancora uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un processo di distensione e di democratizzazione dell'intera area mediorientale, e quindi dell'intero Mediterraneo, e che è causa di innesco di tensioni ulteriori. Si tratta di un conflitto in cui le istituzioni europee ancora non riescono a muoversi in modo uniforme, non hanno assunto un ruolo persuasivo persuasivo nell'incoraggiare la via del dialogo e del negoziato e lasciano tutto in mano all'America. Ecco perché è decisivo l'appuntamento di oggi, per la direzione che, con questa risoluzione, si è voluto tracciare verso un rafforzamento di una diplomazia che possa essere volta alla cooperazione e coinvolga primariamente i popoli degli Stati membri, in modo continuo e permanente. È per tutto questo che si voterà convintamente sì a questa risoluzione.

assolutamente esaustivi e che sposiamo in pieno, vogliamo esprimere intanto vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla 14a Commissione e dai relatori per questa proposta di risoluzione che consideriamo assolutamente importante, utile, positiva e di straordinaria importanza strategica nonché di grande attualità. come ora - secondo noi - è necessario, anche alla luce di quanto è stato detto in precedenza, considerare il nostro Mediterraneo come una macroregione, dove devono essere privilegiati gli interscambi dal punto di vista economico, commerciale ma soprattutto culturale. Lo scambio culturale, soprattutto tra i giovani, l'idea l'idea di un grande Erasmus del nostro Mediterraneo, ci convince e ci attrae, perché - secondo noi - ha una validità assoluta nella crescita e nell'emancipazione culturale, e quindi democratica, di taluni Paesi, soprattutto del Nord Africa, e in particolare della Libia, che è l'anello debole di una potenziale stabilità che noi andiamo a cercare in quell'area. Questa macroregione mediterranea deve condividere con l'Europa caratteristiche, priorità e politiche comuni atte a sviluppare modelli capaci di coinvolgere non solo i Governi ma anche la società civile, garantendo, quindi, percorsi di democratizzazione ed emancipazione culturale - come dicevo - dei Paesi nordafricani che si affacciano sul Mediterraneo, la cui interlocuzione e dialogo sono fondamentali. Così come sono fondamentali programmi finalizzati alla riduzione della povertà e del malessere presenti nelle zone interessate; malessere che contribuisce alla instabilità politica, al terrorismo e al fenomeno dei flussi migratori. Su questo tema, chiaramente, riteniamo di discostarci

ripartendo le responsabilità e gli impegni tra tutti gli Stati membri, non limitandosi ad intervenire solo in situazioni di emergenza ma affrontando a monte la causa del fenomeno. Ecco, quindi, il ruolo dell'Europa nella macroregione mediterranea, nella stabilizzazione e nella democratizzazione dei Paesi nordafricani, in particolare dicevamo prima - la Libia. Il modello chiaramente è quello della Tunisia, che costituisce un riferimento positivo ed un esempio per tutti gli altri Paesi del Mediterraneo, e ne abbiamo avuto prova

alle Camere sulla politica mediterranea dell'Unione europea e propone l'istituzione di una sessione parlamentare annuale legata alle tematiche del Mediterraneo, così da coinvolgere ed informare sempre il Parlamento.

bisognerebbe riflettere, visto che abbiamo in ballo il decreto antiterrorismo e tante altre norme che dovremo votare nei prossimi giorni. Eppure, oggi,

Senatore Crimi, ovviamente la Presidenza e tutto il Senato si associano al cordoglio. Le notizie - com'è noto - sono ancora molto frammentarie, ma credo che la riflessione si svolgerà nei tempi giusti. Nel frattempo, la Presidenza è già in contatto con il Governo

Le comuni ed indissolubili matrici storiche e culturali danno vita a quella che è stata più volte denominata la regione euromediterranea: è per questo che l'equilibrio politico e sociale dell'area delle sponde del Sud del Mediterraneo è di primaria importanza. Stabilizzare i Paesi della cosiddetta primavera araba vuol dire frenare l'immigrazione, soprattutto clandestina, e la tratta di esseri umani. È perciò importante l'impegno di permettere la presentazione della richiesta di asilo nei Paesi di origine e quello di rivedere la regolamentazione europea sull'immigrazione, come da sempre richiesto dal Gruppo Movimento 5 Stelle e come proposto anche da un nostro disegno di legge, che l'attualità impone di discutere tutti insieme, senza bandiere né barriere. Noi siamo pronti: la situazione contingente impone provvedimenti fattivi. Non limitiamoci, come al solito, a mettere delle toppe e a fare la parte dei riparatori, quando invece è ora di costruire e di prevenire. Dobbiamo dare una seria sferzata al fenomeno delle tratte, alla gestione criminosa dei barconi della speranza, e dobbiamo dare e ridare dignità all'essere umano. votare una risoluzione più che mai opportuna, che però dovrà avere un seguito reale e non rimanere in queste stanze. Il bacino del Mediterraneo ha un'importanza strategica, sotto tutti punti di vista: commerciali, sociali e politici. Il ruolo dell'Italia potrà essere quello di protagonista o addirittura di capofila per lo sviluppo di questo bacino, in una visione proficua. Basti pensare alle potenzialità commerciali, a quelle agricole e a quelle alimentari, che oggi sono invece impostate più in chiave concorrenziale, spesso scorretta e senza il controllo delle produzioni che arrivano da noi, dando talvolta ai Paesi del Nord Africa un ruolo di crocevia per le produzioni intensive e geneticamente modificate - come ad esempio quelle del Brasile - dirette ai grandi mercati di Cina e Russia. muovendo in direzione contraria rispetto ai buoni propositi presenti nel testo in esame: l'IMU agricola e l'Expo, sponsorizzato dalle multinazionali dell'alimentazione, come la nota catena americana, danno poco spolvero alle nostre eccellenze e alle potenzialità della area mediterranea. E noi oggi subiamo inermi. La situazione della Libia deve essere risolta a livello diplomatico ed eventuali azioni europee devono puntare alla cooperazione e allo sviluppo, soprattutto con l'impiego di forze civili. Anche in questo caso il fenomeno va stroncato all'origine, ovvero alla radice, corsa al profitto a tutti i costi e sulla strumentalizzazione della religione. Il rubinetto della produzione e della fornitura di armi deve essere chiuso. I pretesti per la guerriglia, che si schermano dietro ad una pseudovisione religiosa, devono essere ridotti a zero. L'azione diplomatica deve essere seria e di uno spessore tale da non consentire più pasticci, perché si tratta di un vero e proprio *pot-pourri* di errori consecutivi, caso della questione palestinese, che oggi rischia di mettere un intero popolo in ginocchio, anche dal punto di vista umanitario. Guardiamo a quanto sta accadendo nel campo profughi di Yarmuk in Siria, dove ci sono decine di migliaia di persone in condizioni disperate,

un vero inferno nell'inferno, per decine di migliaia di persone, prese nella morsa violenta dello Stato islamico e del Fronte al-Nusra, che oggi pare controllino l'80 per cento Ribadiamo e ripetiamo le nostre domande: chi arma lo Stato islamico? Davvero l'azione diplomatica non ha mai potuto prevenire questo stato di cose? Purtroppo sembra che gli equilibri legati al profitto abbiano il sopravvento sulla dignità umana.

Servono quelle azioni che, dallo scorso novembre, quando votammo il precedente testo, non sono mai state messe in campo. È dunque l'ora di passare dalla parola all'azione: noi siamo pronti. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'esame da parte della nostra Assemblea di questa risoluzione e delle problematiche dell'area del Mediterraneo in genere è un fatto molto positivo, che il Gruppo di Forza Italia saluta con favore, sia per il suo significato politico, sia per una serie di ragioni di ordine fattuale, su cui mi soffermerò brevemente. Anzitutto sul piano politico, un dibattito sul Mediterraneo, cioè sull'area geografica che vede l'Italia in posizione centrale, non solo a livello geografico, ma anche a livello storico, culturale ed economico, è quanto mai importante nell'attuale fase storica in cui purtroppo il *mare nostrum* è scosso da tensioni e violenze che addolorano e fanno riflettere profondamente sulle vicende geopolitiche della regione. È importante, inoltre, che nella risoluzione si parli di Mediterraneo anche da un punto di vista europeo, perché effettivamente - come questa mattina è stato ricordato anche nell'intervento del presidente Casini con il corollario delle poco fortunate iniziative intergovernative, opportunamente richiamate nelle premesse della risoluzione, dal Processo di Barcellona all'Unione per il Mediterraneo - è stata negli ultimi anni assente o, nel migliore dei casi, poco presente rispetto alle vicende, a volte drammatiche, che hanno avuto luogo nel Maghreb e in Medio Oriente. Peraltro, in questa sede non posso non evidenziare come - a nostro parere - anche il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea sia stato, sul piano delle politiche mediterranee a livello comunitario, un'occasione persa: ci sono stati molti proclami, ma pochi fatti. Le vicende a tutti note intorno ai flussi migratori provenienti da un Maghreb, in molti punti devastato dall'instabilità e alcune volte dalla guerra civile, sono emblematiche in questo caso. Certo, apprezziamo che, nella risoluzione al nostro esame, si richiami la necessità di una responsabilità realmente condivisa sulle politiche di controllo e gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Ma, al tempo stesso, non possiamo non sottolineare che da molti, troppi anni vi sono discorsi già tante volte ascoltati ma che poi, nel concreto, non hanno portato a sviluppi realmente positivi. L'Italia subisce un peso insopportabile e gli altri Paesi europei affacciati sul Mediterraneo, pur con flussi e problematiche peculiari, vivono spesso una situazione simile, come evidenziato anche nel passaggio, molto opportuno, sul Gruppo Mediterraneo composto, oltre che da noi, anche da Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia, Malta e Francia. Non vi è dubbio quindi che, tra le priorità da affrontare, abbia carattere di primaria importanza quella relativa ai fenomeni dell'immigrazione e della fuga delle popolazioni civili dai teatri di combattimento: milioni di persone che perdono tutto, strappate dalle proprie radici. Dobbiamo ancora lavorare molto su questo versante, perché è inaccettabile lasciare donne e bambini vivere in queste condizioni disumane - da una parte - e trasformare il Mediterraneo in un letto di morte - dall'altra - a causa del traffico criminale degli immigrati. A questo proposito, il riferimento alle missioni Mare nostrum e Triton è da noi non condiviso, proprio perché sono il segno del fallimento di una politica di contrasto di questo tipo di problema. In definitiva, la risoluzione ci aiuta a riflettere su quello che deve essere il ruolo - anche in tempi nei quali troppe volte questa funzione viene messa in secondo piano di fronte alle azioni dei Governi - del Parlamento: ovvero un ruolo di incontro di idee, di dibattito, di approfondimento ma anche di pungolo, appunto, nei confronti del Governo. Su questo piano desidero sottolineare la funzione davvero importante e troppe volte sottovalutata della cosiddetta diplomazia parlamentare. Nella risoluzione si fa riferimento alla funzione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM). A questo proposito, invito a leggere la la relazione che la Commissione europea ha svolto in questi giorni e che è in pubblicazione, relativa al funzionamento degli organismi internazionali che guardano al Mediterraneo, quale analizza le funzioni dell'APEM in senso critico, ma analizza in senso positivo l'azione di altre organizzazioni. Ecco perché colgo questa preziosa occasione per sottolineare come il Parlamento italiano aderisca anche all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, tra i propri principi, quelli che vengono enunciati in questa risoluzione e che negli ultimi anni (in stretto coordinamento con le Nazioni Unite, in cui siede come osservatore permanente presso l'Assemblea generale) ha fatto molto nella ricerca di canali di dialogo in zone purtroppo colpite da conflitti e guerre, dalla Siria alla Libia, fino alla Terra Santa, e che ha visto l'Italia alla sua Presidenza fino al febbraio scorso e che ora vede un suo rappresentante, la collega Fattorini, sedere in rappresentanza del nostro Parlamento come vice Presidente e Presidente di una Commissione. Vi sono state e vi sono tuttora molte iniziative sui binari della diplomazia parlamentare, che vanno sostenute e fatte conoscere. Ricordo quanto fatto, anche in tempi recentissimi, proprio dall'Assemblea del Mediterraneo, sul contrasto al terrorismo, sul fenomeno gravissimo dei *foreign fighters*. Proprio qui a Roma, il mese scorso, c'è stato un importante incontro tra parlamentari dei Paesi del Maghreb per un corso di formazione, voluto dalle Nazioni Unite e sponsorizzato economicamente dall'Unione europea, per quanto riguarda la funzione legislativa dei Parlamenti in funzione antiterrorismo. sul rilancio del Dialogo 5+5 tra i Paesi del Mediterraneo occidentale, sulla protezione del patrimonio storico-culturale dagli scempi dei terroristi dell'ISIS e sulla formazione degli studenti. Ma anche in campo economico ben fa la risoluzione a richiamare l'idea della banca mediterranea, fatta fallire dalla Germania e dai Paesi del Nord Europa, che non l'hanno mai sostenuta e voluta, fino a costringere l'Italia,

di *partnership* mediterraneo, guardando in modo particolare all'occupazione, allo sviluppo dell'imprenditorialità e al settore delle piccole e medie imprese. Da questo punto di vista noi, come Italia, abbiamo le carte in regola per avere avuto l'intuizione giusta, al contrario di altri. Inoltre, è prioritario, tornando al tema dell'immigrazione, già prima trattato, l'impegno per chiedere una revisione dell'accordo Dublino II, così da assicurare che l'Italia non sia sola nel fronteggiare il flusso migratorio che risulta dai vari teatri di guerra della regione. Desidero cogliere questa occasione per evidenziare che il nostro Parlamento, così come dovrebbe essere per tutti i Parlamenti dei Paesi mediterranei, deve e può essere strumento di una grande diplomazia partecipativa per promuovere, in parallelo ai canali intergovernativi che regolano le grandi vicende geopolitiche di questo nostro tempo così complesso, l'incontro tra società civili e tra i tanti giovani, innanzitutto per riflettere, discutere e creare un vero tessuto di cooperazione e co-sviluppo lungo le direttrici del Mare nostrum. È con questo spirito mi consentirete, con un auspicio che da oggi vi siano altre occasioni per dibattere in Parlamento sul Mediterraneo, cioè sulla casa dell'Italia, che in conclusione

La Presidenza è in costante contatto sia per seguire l'esito che per capire quando il Governo potrà riferire sui fatti. COCIANCICH *(PD)*. Credo che molte cose siano state dette in questo dibattito e credo che sia inutile che io oggi le ripeta.

un'indagine per la quale ringrazio il presidente Chiti e i relatori che hanno offerto la possibilità di un approfondimento reale di tante questioni che

Questo processo di Barcellona è stato via via colpevolmente abbandonato da tutti. Abbiamo sentito il senso di frustrazione degli ambasciatori dei Paesi della riva Sud del Mediterraneo, che si erano impegnati in prima persona. Ricordo, per esempio, l'audizione dell'ambasciatore del Marocco. Questo

E quando non si cura, non si previene, non si anticipano i problemi, poi se ne pagano duramente le conseguenze. Oggi vediamo il grande disastro presente nella sponda Sud del Mediterraneo. Paesi che pochi anni fa salutavamo come all'alba di una nuova primavera sono oggi dilaniati dalla guerra civile, da una guerra che non può essere ricondotta esclusivamente al conflitto israelo-palestinese, come tante volte viene detto. In questo caso è un conflitto che riguarda

tra i fratelli musulmani e coloro che invece non appartengono alla componente più radicale), tra i salafiti e coloro che invece aspirano ad una società

noi abbiamo abbandonato questo dialogo, abbiamo abbandonato questo dibattito e abbiamo lasciato che questi Paesi percorressero la strada in perfetta solitudine. Dobbiamo ricordare che, dopo la Seconda guerra mondiale, nell'Europa occidentale nell'Europa occidentale il grande Piano Marshall ha costituito un fondamento sulla base del quale i nostri popoli hanno potuto ritornare ad una floridezza economica, al pieno godimento dei diritti civili ed economici. Credo che il processo di Barcellona avrebbe potuto rappresentare la premessa per un Piano Marshall che investisse l'area del Mediterraneo nel suo insieme.

sia l'Europa sia l'Italia ad un ruolo sempre più marginale nel nostro mondo. In particolare, se l'Italia non sarà capace di imporre questa agenda - come aveva tentato di fare Sarkozy alcuni anni fa proponendo l'unione del Mediterraneo, salvo poi abbandonare

autocondannerà se stessa ad una marginalità nel dibattito politico. Ben venga quindi una sessione permanente del Parlamento. Credo che il Parlamento debba avere un ruolo centrale, perché questo genere di iniziative non possono essere lasciate esclusivamente al Governo. È necessario che i Parlamenti facciano la loro parte, che la società civile faccia la sua parte, che tutti noi ci si renda protagonisti di questo processo. Non possono essere sempre e soltanto gli altri a prendere l'iniziativa, e la colpa non può essere sempre e soltanto degli altri. Allo stesso modo non ha senso continuare a vedere i rapporti euromediterranei soltanto in termini prevenzione dell'immigrazione illegale. Questo è un tema grave, ma non può essere soltanto questa la risposta. Frontex è stata sicuramente un'iniziativa che ha avuto il merito di coinvolgere l'Unione europea, ma è indubbio che la risposta, a livello europeo, sia ancora insufficiente perché le risorse messe a disposizione non sono adeguate. Noi dobbiamo avere un coinvolgimento non solo simbolico, ma effettivo, il che vuol dire un'attenzione prioritaria di tutta l'Unione europea su questi temi. Concludendo, Presidente, credo veramente che questo lavoro sia stato molto positivo. L'inchiesta che è stata svolta ha messo in evidenza tanti temi, tracce e fili rossi che dovranno essere esplorati

l'Asia, l'Africa e l'Europa. Per questo motivo il Partito Democratico dichiara il voto favorevole a questa risoluzione il mio voto di astensione su questa risoluzione perché la ritengo assolutamente debole e incompleta dinanzi all'importanza del tema che tratta. Basta vedere le premesse: mancano quattro dei punti che hanno dato luogo alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo. Non sono esaminate le questioni ambientali, le questioni energetiche energetiche e le questioni relative al programma di protezione civile. Sono esaminate solamente alcune questioni di convenienza dell'attuale Governo per la sua azione assolutamente debole. Non è prevista una specifica richiesta al Parlamento europeo e alla Commissione europea di inserire, ogni qual volta assume una deliberazione, uno specifico riferimento alle tipicità mediterranee, sia nelle direttive che nelle risoluzioni. quanto riguarda il piano Juncker, alcuna previsione di richiesta di destinazione di una quota di quegli investimenti ad imprese che vanno ad operare a cavallo tra gli interessi europei e gli interessi mediterranei.

questa è la risoluzione del Parlamento italiano sul Mediterraneo, allora io credo che altro che i vent'anni che ci separano da Barcellona o gli otto che ci separano dalla fondazione dell'Unione per il Mediterraneo; molti decenni passeranno ancora prima che si ottenga una vera politica mediterranea. Non si parla di turismo, non si parla di agricoltura e di tutte quelle risorse che il Mediterraneo dovrebbe avere e mettere a disposizione delle sue popolazioni per poter crescere. La visione internazionale, dal punto di vista delle criticità, si limita a trattare il caso della Libia e del conflitto israelo-palestinese e volutamente ignora la questione cipriota, la questione yemenita e la stessa questione del Mar Nero perché il Mediterraneo non è solo una espressione geografica, come altri in passato hanno detto per l'Italia, ma è un'area di interesse complessiva, Non si prende in considerazione la nuova politica dei trasporti che dovrebbe essere sin da ora prevista dopo il nuovo taglio di Suez, non si entra nel merito di tantissime questioni che dovrebbero essere affrontate con maggiore determinazione dal Paese che è maggiormente interessato allo sviluppo del Mediterraneo. che in futuro si possano avere decisioni molto più incisive sulla nostra posizione nei confronti di ciò che in Europa accade. Un'Europa sempre continentale, sempre proiettata al Nord e all'Est e sempre distratta e disattenta rispetto a quanto accade nel Mediterraneo. colleghi, le notizie che giungono da Milano confermano che i morti sono tre mentre un'altra persona sta lottando tra la vita e la morte.

minuto di silenzio).* Confermo che continueremo a restare in contatto con il Governo affinché, appena possibile, aggiorni il Senato sugli avvenimenti, che ovviamente suscitano grandissima preoccupazione ed enormi interrogativi.

colleghi, il nuovo piano di razionalizzazione varato da Poste italiane lo scorso dicembre prevede a livello nazionale la chiusura di ben 455 uffici postali e l'apertura a giorni alterni di altri 608, ritenuti improduttivi o diseconomici. Nella mia Regione, la Lombardia, è prevista la chiusura di 65 uffici e la riduzione dell'orario di apertura in altri 120. Per calarci nel mondo reale, che troppo spesso è dimenticato da chi prende le decisioni, e solo per fare qualche esempio, è prevista la chiusura degli uffici delle frazioni di Malnate, Cairate, Gazzada Schianno e di Luino in provincia di Varese dell'ufficio postale della frazione di Gallignano, che dista ben 6 chilometri dal comune di Soncino nel cremonese. Nel lecchese, sono destinati alla chiusura sette uffici in frazioni, tra cui Sala al Barro e Rossino, che appartengono a Comuni montani. In provincia di Sondrio, definita interamente montana, la scure sta invece per abbattersi a Madonna di Tirano e a Cosio Stazione. La decisione di Poste è da condannare nel metodo e nel merito; perché il piano è stato assunto unilateralmente, senza coinvolgere i Comuni interessati, i quali solo a fine gennaio hanno appreso la notizia dalla stampa e da fonti sindacali, diverse settimane prima della comunicazione ufficiale; nel merito, perché molti uffici colpiti si trovano in frazioni periferiche o in frazioni di Comuni montani che in questi anni stanno vedendo scomparire scuole, negozi, studi medici, farmacie. Questo è un colpo mortale alla vita sociale di quelle comunità, è un contributo allo spopolamento dei territori. Questo, dopo l'IVA sul pellet, le minori agevolazioni sul gasolio per riscaldamento e l'IMU sugli impianti a fune è un'altra dura batosta alla montagna. Il piano di Poste italiane che - ricordiamolo - gestisce i servizi in una condizione di sostanziale monopolio, farà precipitare ancor di più la qualità del servizio, rinnegando la *ratio* propria del servizio universale. Le comunità locali coinvolte, le famiglie, le imprese, i sindaci, gli stessi dipendenti di Poste sono allarmati e seriamente preoccupati. Ma in particolare terrorizzati sono gli anziani che, come è noto, non hanno l'auto, e che alla posta vanno a piedi per ritirare la pensione e a pagare i bollettini. Questi saranno costretti a fare diversi chilometri basandosi su un trasporto pubblico locale inefficiente e che risentirà ancora di più dei tagli impartiti dal Governo. È da irresponsabili! Anche perché non può essere definita seria la misura di Poste italiane di dotare i porta lettere di palmari. Molti anziani, lo ricordiamo, non hanno il *bancomat*! Sono quegli anziani che da febbraio 2012 si sono visti rastrellare coattivamente i propri risparmi. Poste italiane prima li ha costretti a non riscuotere più la pensione in contanti e dunque a lasciare i propri risparmi sui libretti postali, e ora li "premia" chiudendogli l'ufficio periferico. Un pessimo affare per loro! Fortunatamente contro il piano di Poste si è registrata una mobilitazione generale. Comuni, Province e Regioni e cittadini con petizioni popolari, hanno reagito con determinazione per tentare di bloccare e far rivedere l'operazione. Anche da parte di molti parlamentari c'è stata mobilitazione, e non solo di quelli della Lega Nord, movimento da sempre attento alle istanze ed esigenze del territorio. Nonostante voci di corridoio parlino di un rinvio di qualche settimana dell'entrata in vigore del piano, che a tutt'oggi risulta ufficialmente previsto per lunedì prossimo 13 aprile, considerata la persistente assenza di risposte dei ministri destinatari di moltissime interrogazioni parlamentari, come Carroccio abbiamo ritenuto opportuno che l'Assemblea del Senato si esprimesse su questa mozione, presentata il 3 marzo (oltre un mese fa) per chiedere al Governo di impegnarsi sul problema. Colleghi, pur nella consapevolezza che nell'ottica della *spending review* debba essere operata una razionalizzazione delle poste, accompagnata ad uno sviluppo dei servizi innovativi, questa è l'occasione per dimostrare, con i fatti e non con interrogazioni - che, ahimé, finiscono sempre su un binario morto - che siamo tutti per la tutela dei territori deboli. Citando il detto: «A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca», non vorremmo che lo *stop* al piano ufficioso sia tattico e motivato motivato dalle elezioni amministrative alle porte. Non ci rassicurano, infatti, le lettere di disdetta inviate già nei giorni scorsi da Poste ai proprietari dei locali dove è in affitto l'ufficio candidato alla chiusura. vengo, dunque, agli impegni che chiediamo al Governo con la nostra mozione: 1) fornire la lista degli uffici postali coinvolti nella razionalizzazione, specificando per ognuno il rapporto tra costi e benefici, i costi delle locazioni, i depositi medi, il numero della popolazione servita; 2) effettuare una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione al fine di valutare di volta in volta la portata dei disagi arrecati all'utenza; 3) pubblicare l'ammontare dei contributi statali erogati negli ultimi cinque anni a Poste italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale; 4) rivedere, valutato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, l'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere, dire ridistribuire i contributi statali e riconsiderare le convenzioni alla luce della razionalizzazione dei servizi offerti; 5) rendere noto l'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione; 6) valutare la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste italiane; 7) intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere normativo - leggasi delibere dell'Agcom affinché venga garantita la permanenza degli uffici postali già presenti nei Comuni rurali o nei Comuni montani, insomma nelle aree svantaggiate; 8) assicurare un 8) assicurare un rinvio dell'entrata in vigore del piano di razionalizzazione, ciò per consentire una concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale. Colleghi, quelle che ho in mano sono le tante interrogazioni che dalla fine di gennaio ad oggi sono state depositate per denunciare il problema. Sono presentate da tutti partiti e sottoscritte da moltissimi di voi. Farei certamente prima a citare coloro che non compaiono in questi documenti, intendiamoci, non per additarli, ma proprio per sottolineare - sono certo - la convinta e trasversale preoccupazione che il piano di Poste sta determinando. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. I senatori della Lega, di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle, del Gruppo Misto, di quello delle Autonomie e certamente anche quelli del segnalano qui il problema generale e citano i tanti Comuni italiani di tutte le Regioni - ripeto, tutte le Regioni - su cui dovrebbe abbattersi la scure di Poste italiane. Tutti sostanzialmente chiedono due cose: la sospensione del piano e la revisione concertata dei criteri per la tutela delle aree svantaggiate. Ebbene, la nostra mozione va incisivamente proprio in quella direzione ed è per questo che confidiamo possa essere sostenuta.

Poste italiane SpA, fondata nel 1862, è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100 per cento dallo Stato italiano tramite il Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo gli ultimi dati finanziari disponibili, relativi al 2013, essa conta ricavi per 8,978 miliardi di euro ed un utile netto di 708 milioni, mentre il gruppo Poste italiane, nel cui bilancio consolidato incidono circa 25 società da questo controllate - inclusa Poste italiane - vede ricavi di esercizio per 26,268 miliardi ed un utile netto che sopravanza i 1.000 milioni. Va rilevato che la maggior parte dei ricavi viene effettuata nelle sedi fisiche dei circa 13.000 uffici postali distribuiti in tutta Italia, dove vengono realizzate circa 50 milioni di operazioni al giorno. Vorrei fornirvi qualche dato 6 milioni di conti correnti postali, 13 milioni di carte prepagate Postepay (pari a circa il 25 per cento del mercato delle carte prepagate), 6,8 milioni di carte Postamat, 13 milioni di invii postali al giorno, 220.000 pacchi pacchi giornalieri, 30 milioni di bollettini al mese, 250 milioni di raccomandate l'anno. In data 16 dicembre 2014, l'ingegner Francesco Caio, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Poste italiane, ha presentato il nuovo piano strategico a cinque anni, denominato «Poste 2020». Nel piano è prevista la progressiva chiusura di 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura di ulteriori 600, ritenuti improduttivi, nonché antieconomici. Da questa decisione si evince che il *business plan* messo in atto da Poste italiane dà preminenza ad una politica del profitto derivante dal *business* dei servizi di assicurazione, dei servizi bancari e finanziari, delle carte di credito e ricaricabili e della telefonia cellulare, a discapito delle reali necessità della popolazione, che necessita della fornitura di servizi di prossimità, anche in condizione di probabile mancata redditività. I servizi postali sono di vitale importanza per l'esecuzione di tantissime attività quotidiane, quali il prelievo di contante per i titolari di conti correnti postali, il pagamento delle utenze, il deposito di valuta nei libretti postali al portatore, l'invio di comunicazioni urgenti. La paventata chiusura o la limitazione degli orari degli uffici postali pone in gravi difficoltà cittadini ed aziende. In particolare nei piccoli Comuni, specialmente in quelli montani, la soppressione di un ufficio postale, al pari di un presidio medico o di uno sportello bancario, rappresenterebbe il venir meno di un servizio essenziale per una comunità; penso, in modo particolare, ai cittadini anziani o diversamente abili. una reale quanto imprescindibile necessità di orientare la gestione dei servizi alla sostenibilità economica, ma ciò non deve avvenire a discapito del servizio e del mantenimento dei presidi sul territorio. Il presupposto che il risparmio postale goda della garanzia dello Stato fin dal 1875 fa in modo che presso gli uffici postali risultino depositati circa 320 miliardi È quindi evidente che la garanzia dello Stato sul risparmio postale inviti i cittadini ad affidare i propri risparmi ad un soggetto, Poste italiane, che offre maggiori garanzie rispetto ad ogni altro operatore bancario. In sostanza, il gruppo Poste Italiane è una realtà che si confronta con il mercato italiano del risparmio e dei servizi ad esso inerenti in una posizione di estremo privilegio, che è ancora più accentuato dal fatto di essere una società per azioni a controllo pubblico.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo opportuno formulare queste considerazioni. In primo luogo, l'eventuale privatizzazione totale dell'azienda o la soppressione del servizio a livello locale non possono essere trattati unilateralmente dall'azienda o dal Governo, ma devono tenere invece conto di una discussione da effettuare a livello Su questa base, si invita il gruppo Poste italiane alla redazione di un nuovo piano industriale per gli anni 2015-2019 solamente dopo aver reso pubbliche le *performance* complessive degli uffici ed aver misurato i disagi arrecati alle famiglie e alle aziende che deriverebbero dalla chiusura di alcuni uffici postali. il Governo a valutare la possibilità di verificare il piano succitato coinvolgendo anche l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), per stabilire quali siano gli sportelli da ritenere comunque indispensabili, anche tenendo conto del processo di aggregazione dei piccoli Comuni. a rendere noti i criteri oggettivi ed omogenei che giustificherebbero l'intenzione di chiudere o ridimensionare gli orari di apertura degli uffici postali, attraverso una concertazione tra la direzione di Poste italiane SpA e gli amministratori locali, per evitare che decisioni unilaterali arrechino disagi agli abitanti delle comunità rurali del Paese, che si vedrebbero privati dell'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, così come previsto finora dall'accordo siglato tra Poste italiane e lo Stato. ad attuare interventi per far sì che Poste italiane SpA si occupi e garantisca pienamente il servizio pubblico essenziale che presuppone la prossimità e la copertura del territorio nazionale anche per meglio fornire, come accade già in logica di mercato, gli altri servizi connessi. Il nostro auspicio è dare attuazione ai punti precedentemente esposti del collocamento della quota minoritaria del 40 per cento delle azioni di Poste italiane sul mercato regolamentare. regolamentare. Questo è un tema trasversale su cui tanti parlamentari hanno manifestato la propria intenzione e credo che la nostra mozione possa raccogliere il consenso dell'Assemblea proprio perché va nel senso dell'organizzazione fondamentale di questo Paese; un Paese che si basa sulla prossimità e su servizi importanti come quello che la posta rende ai cittadini tutti i giorni. È per questo che confidiamo in una votazione favorevole alla nostra mozione.

sarà abbastanza breve, anche in ragione del fatto che molte delle questioni che sono state oggetto della nostra mozione sono contenute nelle illustrazioni che hanno preceduto questo mio intervento. Siamo di fronte ad un ennesimo percorso di cosiddetta razionalizzazione dei servizi, dove «razionalizzazione» sta per ridimensionamento, smantellamento, riduzione di diritti. Lo dico perché il servizio postale universale è concepito, nelle leggi come nei trattati internazionali, come un diritto da tutelare e un servizio da garantire anche nelle realtà più decentrate e periferiche del Paese.

assolutamente come un diritto il cui esercizio va tutelato, anche ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione.

che più di ogni altra utilizza quel tipo di servizio, e pongono problemi di sicurezza. Le ipotesi di sostituire quell'attività con il cosiddetto portalettere telematico problemi di sicurezza da non sottovalutare, proprio per la popolazione anziana che è interessata a questo servizio, non solo per le questioni di corrispondenza privata, ma anche per l'utilizzo dei servizi finanziari che sono garantiti dalle poste. C'è un problema di relazione con il sistema delle autonomie locali; questo piano deve essere condiviso

che lede i diritti di una popolazione in modo assolutamente intollerabile sotto il profilo del rispetto dei principi di uguaglianza contenuti nella Costituzione. In Sardegna viene ridimensionata notevolmente la presenza delle Poste e vengono colpiti Cortoghiana del Sulcis, trova in prossimità della miniera di Nuraxi Figus, Turri, Genuri, Tuili, Pauli Arbarei, Nurallao, Borutta, Esporlatu, Ozieri, Nughedu San Nicolò, Ardara e Romana, tutti piccoli Comuni

Ecco perché era ed è prevista nella procedura che si tenga conto dell'opinione degli enti locali, cosa che invece è stata fatta in modo molto superficiale ed insoddisfacente.

ovvero l'Agcom, che deve esercitare questa funzione mantenendo quei livelli di di ramificazione del servizio postale che fino ad oggi almeno sono stati garantiti (parlo del 96 per cento Detto questo, penso vi sia la possibilità di concludere positivamente la discussione delle mozioni presentate, anche approvando

cose che dovrebbero essere garantite senza bisogno dell'intervento dell'Aula parlamentare, ma che purtroppo non lo sono state. In sollecitare Agcom e Poste italiane affinché venga pubblicata quanto prima la lista completa degli uffici postali oggetto di razionalizzazione, al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo in capo al fornitore del servizio universale

chiediamo a Poste italiane di mantenere la sospensione dell'attuazione del piano di razionalizzazione, così com'è stato predisposto, per garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, affinché possa verificarsi l'effettivo rispetto delle esigenze dei cittadini e della specificità di tutti i territori interessati. individuate soluzioni che compensino concretamente i disagi legati all'eventuale chiusura di sportelli o riduzione di orario che dovessero derivare da

chiarisca in modo preciso l'utilizzo del cosiddetto portalettere telematico, per capire quale incidenza avrebbe questo strumento soprattutto sulla serenità e sull'operatività sull'accesso all'operatività del servizio da parte della nostra popolazione anziana.

Esso prevede, tra le altre, la chiusura di oltre 450 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in 608 uffici. La riorganizzazione prevista nel Piano in questione preoccupa moltissimo per le sue ricadute sociali, considerato che Poste Italiane è tenuta a garantire l'espletamento di un servizio di particolare valore sociale, anche in forza di un contratto di programma stipulato con il Governo.

per consentire un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e per individuare possibili soluzioni alternative. Si pone quindi con molta forza l'esigenza di rendere socialmente sostenibile il piano di Poste italiane. Infatti i servizi postali rappresentano un servizio imprescindibile per lo svolgimento delle attività quotidiane delle famiglie e delle imprese, come ben sappiamo. Questa riorganizzazione contenuta nel Piano, se non verrà riconsiderata, determinerebbe disservizi ai cittadini, in special modo a quelli appartenenti alle fasce più deboli, come gli anziani o le persone con ridotta mobilità. Va inoltre sottolineato come il Piano presentato colpirebbe in particolare gli uffici postali nelle piccole realtà, soprattutto collinari e montane, anche se ricomprese nei Comuni di pianura.

Infine, va considerato che il Governo, con l'approvazione dell'ordine del giorno del 30 novembre 2014, si è impegnato a considerare ogni atto di competenza finalizzato ad assicurare, durante l'*iter* di privatizzazione di Poste italiane SpA, la tutela, la protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali attuali di tutti i lavoratori impiegati presso la società, con particolare riferimento a quelli operanti proprio nel settore del recapito postale. mozione, il Partito Democratico intende quindi impegnare il Governo, nella sua qualità di garante e responsabile del servizio postale nazionale, a rinviare innanzitutto l'entrata in vigore del piano di di razionalizzazione di Poste, a considerare con particolare attenzione l'impatto sociale che tale piano produrrebbe sulle singole realtà locali interessate dalla riorganizzazione, ad intervenire su Poste italiane SpA, per favorire una revisione del piano di riorganizzazione degli uffici postali che tenga conto delle specificità del contesto sociale ed economico, dell'insediamento abitativo, dell'inclusione sociale per le categorie che abbiamo ricordato, delle condizioni particolari in cui versano i Comuni interessati, con attenzione alle aree pedemontane, caratterizzate da località, frazioni collinari o montane isolate, anche se ricomprese in Comuni di pianura. Si impegna dunque ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché Poste italiane SpA proceda all'elaborazione di un Piano che preveda la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti dalla riorganizzazione, i diversi livelli istituzionali, nazionali e regionali, coinvolgendo le realtà territoriali nella valutazione delle situazioni situazioni più rilevanti e al contempo verificando concretamente possibili soluzioni alternative che possano attenuare gli effetti negativi della prevista riorganizzazione;

Signora Presidente, colleghi, Governo, ho ascoltato con molto interesse il dibattito su queste mozioni da noi presentate oggi e vorrei sottolineare che secondo me quello che non sta emergendo da questa discussione è il dato politico,

nei giorni scorsi addirittura la Commissione europea è intervenuta pesantemente sul piano perché ne ha di fatto già bocciato una parte che dovrebbe entrare in vigore lunedì prossimo, in particolare la parte che prevede la consegna della posta a giorni alterni, perché viola il diritto di accesso al servizio di posta universale che prevede invece la consegna quotidiana. Da ultimo, secondo me è bene ricordare le parole dell'amministratore delegato di Poste italiane, Caio, il quale ha detto che è comunque disponibile ad intraprendere iniziative di condivisione sul territorio,

come tutti hanno ricordato, prevede un allontanamento da quei criteri di responsabilità sociale che sono addirittura citati nello statuto e nel codice etico di Poste italiane o se vogliamo avvicinarci a questi criteri. È chiaro che Poste italiane nasce con una *mission* ben inquadrata e specifica. Da questa *mission* nel tempo ci siamo allontanati.

a garanzia delle zone svantaggiate, rurali, montane e delle isole minori. Bisogna tener conto delle distanze, della geografia del nostro territorio, che è molto diffuso e non accentrato su pochi centri urbani. Chiediamo che sia garantita l'accessibilità ai servizi postali a tutte le categorie sociali, non solo alle persone che hanno possibilità maggiori, ma soprattutto alle persone disagiate.

potrebbero essere enormemente svantaggiate. Ricordiamo che nella legge denominata salva Italia fu prevista l'obbligatorietà di versamento delle pensioni in conti postali o conti correnti Questo ha vincolato di fatto tutta una serie di persone, un numero molto importante, ad accedere a questi uffici. Dobbiamo tenere in considerazione anche questo aspetto. Chiediamo, inoltre e non da ultimo, la salvaguardia delle condizioni occupazionali. Il piano che prevede lo stralcio di 400 uffici e la riduzione dell'orario di 600 altri uffici porta con sé delle criticità a livello occupazionale. Chiediamo, inoltre, al Governo che vengano prese in considerazione le rilevazioni fatte dalla CONSOB riguardo alla tipologia di servizi offerti e, soprattutto, sul fatto che possa essere presa in considerazione a non esclusività della fornitura di alcuni servizi da parte di Poste. Ciò la mette in una condizione di dominio sul mercato. mercato. Come ultimo punto, come sempre, chiediamo che il Parlamento sia correttamente informato sul piano e su quali sono le modalità di implementazione che l'azienda Poste italiane SpA ha in mente di porre in essere.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, prendo la parola per illustrare l'ordine del giorno con il quale, assieme al collega Berger, chiedo l'impegno del Governo affinché il nuovo piano di riordino di Poste italiane non penalizzi territori già svantaggiati, a cominciare da quelli di montagna. Sul piano di riordino, nelle scorse settimane, non sono mancate le proteste da parte delle comunità interessate e continue sollecitazioni da parte degli enti locali e dei rappresentanti istituzionali, proteste di cui io e altri colleghi ci siamo fatti portavoce. Il consiglio della Provincia autonoma di Trento, ad esempio, ha approvato il 5 marzo scorso una specifica mozione. Alla Camera è stata presentata un'interrogazione promossa dal Gruppo interparlamentare per lo sviluppo della montagna e sottoscritta da ben 55 deputati. Anche in Senato sono state depositate diverse interrogazioni, anche dal sottoscritto, dai colleghi del Gruppo per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, a conferma del fatto che c'è forte preoccupazione sul piano di riordino. Poste Italiane - è stato detto - è una società a capitale interamente pubblico che opera in un regime di sostanziale monopolio ed è naturalmente finanziata dallo Stato. Quindi, ha il dovere di escogitare soluzioni affinché la razionalizzazione del servizio non si prefiguri come cancellazione per specifici territori. È un dovere, questo, regolato anche da specifiche norme, ad iniziare dalla delibera Agcom, che obbliga Poste italiane a confrontarsi con le istituzioni locali con l'obiettivo di limitare al massimo i possibili disagi per le popolazioni interessate, individuando soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale. Il 22 gennaio

di quegli uffici che servono gli utenti che abitano nelle zone remote del Paese, ritenendo prevalente l'esigenza di garantire la fruizione del servizio nelle zone disagiate, anche a fronte di volumi di traffico molto bassi molto bassi e di alti costi di esercizio. Sempre in tale missiva, il garante esplicita chiaramente come i divieti di chiusura - è bene sottolinearlo - tutelano situazioni individuate

la sospensione del piano da parte di Poste italiane per aprire il tavolo di confronto con gli enti locali, in sostanza con le Regioni e le Province autonome. Voglio anche rimarcare che le piccole comunità di montagna hanno saputo negli anni trovare forme di collaborazione con Poste italiane e spesso sono riuscite a risolvere il problema; cito, ad esempio, ad esempio, il caso del Comune di Valfioriana, in Trentino, un territorio costituito da innumerevoli piccolissime frazioni all'inizio della Val di Fiemme, che ha messo a disposizione delle Poste il centro anziani ed ha trovato la formula per collaborare direttamente all'apertura dello sportello. In Trentino si sta anche attivando il mondo della cooperazione

che servono territori a bassa densità abitativa, ma che sono inseriti in un'area particolarmente estesa e con una popolazione tendenzialmente anziana, si configurerebbe come sostanziale cancellazione del servizio. chi conosce la montagna sa bene che il suo spopolamento e il suo impoverimento passano proprio da dinamiche di questo tipo, ovvero dalla difficoltà di chi vi abita ad accedere ai servizi. È, in sostanza, una vicenda che va inserita in una logica più ampia e cioè quella della tutela e valorizzazione

alla rete postale siano effettivamente quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 ottobre del 2008 e che, in particolare, vi sia un intervento nei confronti di Poste italiane affinché coinvolga direttamente nelle scelte gli enti locali interessati e tenga in considerazione le loro proposte. Ma chiediamo anche che si tengano in dovuta considerazione le indicazioni del Gruppo interparlamentare per lo sviluppo della montagna, impedendo che la riorganizzazione del servizio postale si configuri come un concreto impoverimento di comunità, come quello delle zone montane e delle isole minori, già di per sé fortemente penalizzate. Mi rendo conto che i conti devono tornare e che il piano deve rispondere, giustamente, a principi di sostenibilità economica ma sono anche convinto che i risparmi possono essere fatti in altro modo e che quando i territori si spopolano le conseguenze diventano irreversibili. Condivido molte delle considerazioni svolte da chi mi ha preceduto e che hanno rimarcato alcune delle problematiche che ho evidenziato nel nostro ordine del giorno. Mi auguro che il Governo accolga tale ordine del giorno o che l'Aula esprima il suo voto favorevole per evitare una ulteriore penalizzazione di territori che sono già in forte difficoltà.

che si troverebbe a dover subire una ulteriore difficoltà, un ulteriore taglio, a fronte di un sistema di servizi che già, per certi versi, in alcune zone è carente. Quindi questo sostanziale monopolio diventa un disagio, un atto d'imperio, un atto di mancato confronto con i territori e gli enti locali. Pensiamo alle amministrazioni e ai sindaci che sono diventati solo ed unicamente gabellieri per questo Governo che poi non si pone il problema di dare risposte sui servizi. Ed ecco che ancora una volta il Parlamento deve interagire per portare all'attenzione del Governo un problema che è di vitale importanza e di buon senso: senso: bisogna evitare questa interlocuzione ma agire direttamente su quello che, lo ripetiamo, è un servizio dovuto ad alcune aree in particolare, ad alcune situazioni e ad alcune categorie. Ricordiamoci che abbiamo ancora delle grandi realtà con persone anziane alle quali, tra l'altro, una normativa ha imposto di doversi rivolgere agli uffici postali per poter ritirare o depositare le loro pensioni. Quindi è una beffa nella beffa

bocca. Stiamo parlando di cose senza senso, di cose che chi non prova non sa nemmeno capire. Con il nostro ordine del giorno chiediamo, quindi, che sia valutata tutta questa situazione di tagli ai servizi con i territori

devono essere coloro che conoscono la realtà, il territorio, le famiglie, le persone e i servizi necessari. Nessuno nega che ci sia bisogno di arrivare a vedere risparmi anche da tesaurizzare ma concertandoli con i territori, in base anche alle virtuosità

Anche la delibera dell'Agcom fa riferimento a queste aree svantaggiate. È bene evidenziato come le aree a carattere prevalentemente montano o le aree che hanno scarsa densità abitativa

perché Poste italiane faccia riferimento a un servizio come servizio universale e non a un servizio che si basi solo sulla economicità e, quindi, sulle risposte dal punto di vista di risultati aziendali, ma abbia ancora quella natura che tale servizio deve avere.

appunto condivisa e coniugarsi alle esigenze che hanno natura economica ma in particolare, e prima di tutto, natura di servizio per l'utenza che deve accedervi. Con l'ordine del giorno G2 chiediamo tutto questo e siamo certi, vista anche la condivisione sia delle mozioni che degli ordini del giorno (che vanno tutti in questa direzione di un forte rientro di questo taglio senza alcun

vorrei rimanesse agli atti la contezza, che diventa un patrimonio comune, che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, negli ultimi anni è stato interessato da trasformazioni profonde. Non è il momento dell'analisi. Mi limito a citare il cambiamento più importante, il passaggio delle funzioni di regolamentazioni e vigilanza e vigilanza da questo Ministero all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per effetto del decreto legge n. 201 del 2011, poi convertito. Il contratto di programma vigente prescrive che Poste SpA trasmetta all'Autorità, con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e che l'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolga

razionalizzazione risultano essere pienamente rispettosi della normativa vigente. Tuttavia, nonostante questi cambiamenti e le competenze ricordate che rimandano all'Autorità, il Governo non ha ritenuto

Per questo abbiamo promosso un incontro con il presidente di Agcom Cardani e con l'amministratore delegato Caio sollecitato Poste a che l'attuazione del piano fosse preceduta da un confronto serio con le Regioni, i comuni e gli enti locali interessati, non tanto per mera esigenza informativa, quanto perché dal confronto scaturisse la possibilità di trovare insieme soluzioni che riducessero l'impatto sociale di cui ho detto su molti territori, senza compromettere la ricerca di efficienza.

delle realtà coinvolte affinché siano parte attiva nel confronto tra le Regioni e Poste. Non si tratta infatti di un passaggio burocratico. In ogni circostanza, il Ministero ed il Governo complessivamente sono intervenuti per offrire la propria disponibilità ad essere parte attiva e cercare una sintesi tra le esigenze della comunità e quelle dell'azienda. A me è sembrato, sinceramente, che questo spirito

su tutta la parte che riguarda le presmesse, perché se entrassimo nella valutazione delle premesse e della lettura che legittimamente ciascun Gruppo dà del piano e delle sue motivazioni, probabilmente perderemmo la possibilità di accogliere molti degli spunti emersi, mentre credo sia utile che ci siano voci che testimoniano come il Parlamento entri in queste dinamiche e sia capace di farsi carico delle attese.

confronto in atto con gli enti locali, la lista completa degli uffici postali prossimi alla chiusura o interessati da una riduzione dell'orario di apertura, al fine di assicurare il rispetto degli obbilghi in capo al fornitore del servizio universale quale, in particolare, il mantenimento dell'operatività di un ufficio postale nel 96 per cento dei Comuni italiani;**

politico e di relazione tra le amministrazioni locali e Poste per andare oltre i soli criteri del servizio universale: questa è la strada che dobbiamo percorrere.

si impegnasse il Governo a sollecitare l'Agcom alla verifica di ogni misura di razionalizzazione, anche se oggettivamente credo che l'Autorità sia già

«a fornire al Parlamento l'indicazione complessiva dei contributi statali erogati negli ultimi cinque anni a Poste italiane SpA per l'espletamento del servizio pubblico universale».

comma 274, lettera *b),* della legge n. 190 del 2014, ha già rivisto al ribasso l'importo massimo dei trasferimenti a carico della finanza pubblica per lo svolgimento del servizio universale

che più che nostro è della Banca d'Italia, per cui i criteri, i principi e le modalità sono regolati dalla Banca d'Italia

per le eccezioni che quella direttiva ammetteva (le notifiche di atti giudiziari e le violazioni del codice della strada), il Governo,

(sempre perché c'è un rispetto delle prerogative e dei ruoli che non riguardano il Governo). Il punto 8) del dispositivo, che credo

Poste italiane; dunque credo che possa essere accolta la richiesta di vigilare perché sia confermato questo differimento, che noi riteniamo opportuno e che va nel senso dell'impegno chiesto per una fase di concertazione non formale con gli enti locali.

«a verificare che sia confermato il differimento comunicato da Poste» è lo stesso principio della mozione precedente - «fino al termine del confronto in atto con Regioni ed enti locali».

riformulazione: «a sollecitare la società Poste italiane SpA ed ANCI a continuare il confronto costruttivo già in corso, finalizzato a discutere il piano di razionalizzazione degli uffici postali».

arrechino disagi agli abitanti dei Comuni più disagiati del Paese, che si vedrebbero privati dell'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, così come previsto dall'accordo siglato tra le Poste italiane e lo Stato».

ad attuare interventi per far sì che Poste italiane SpA si occupi e garantisca pienamente il servizio pubblico essenziale che presuppone la prossimità e la copertura del territorio nazionale anche per meglio fornire, come accade già in logica di mercato, gli altri servizi

affinché, al termine del confronto in atto con Regioni e Comuni, venga pubblicata la lista completa degli uffici postali prossimi alla chiusura o interessati da una riduzione dell'orario di apertura». Su questo tema mi preme essere chiaro con il Senato.

è mio convincimento che il confronto con gli enti locali possa portare ad una diminuzione del numero degli uffici poi interessati dalla chiusura. obbligano prima Poste a motivare le chiusure annunciate sarà molto più difficile poi per Poste, a mio avviso, ritornare su una decisione che ha motivato pubblicamente, mentre se lo facciamo al termine del confronto credo che facciamo una cosa utile. Esprimo parere Da questo punto di vista condividiamo anche l'esigenza che siano pienamente illustrate e diffuse le opportunità dei nuovi servizi telematici.

a valutare con particolare attenzione l'impatto sociale che il piano di razionalizzazione degli uffici di Poste italiane SpA per gli anni 2015-2019 sollecitando ulteriormente Poste italiane SpA affinché, nel confronto in atto con i diversi livelli istituzionali, ponga particolare attenzione alla necessità di garantire il servizio nelle situazioni più critiche con particolare attenzione alle aree pedemontane caratterizzate dalla presenza di località o frazioni collinari e/o montane isolate ricomprese in comuni di pianura e alle comunità di cittadini in prevalenza anziani a ridotta mobilità;

ad intervenire presso Poste italiane SpA per chiedere che continui a confrontarsi con gli enti locali , al fine di mitigare l'effetto del proprio piano industriale sui servizi offerti, anche a seguito di precedenti interventi di razionalizzazione, garantendo la piena operatività del servizio universale, in particolare modo per i cittadini che risiedono in aree svantaggiate del Paese e/o minore mobilità in considerazione anche dell'età anagrafica; a fare in modo, in particolare, che Poste italiane SpA, anche attraverso impegni programmatici assunti nell'ambito del nuovo contratto adotti iniziative tese a valorizzare la rete capillare degli uffici postali, ed in particolare le potenzialità e le caratteristiche degli stessi quali uffici di prossimità al servizio degli utenti, specialmente negli ambiti territoriali con scarsa densità abitativa e a consetire che gli stessi uffici, in aggiunta alla piena fornitura del servizio postale universale, postale universale, possano fornire - oltre a quanto previsto dal decreto "salva Italia" relativamente al versamento delle pensioni - ulteriori servizi di pubblica utilità al cittadino sulla base di convenzioni con singole pubbliche amministrazioni;

Poste, sollecitata nella definizione di una risposta, comunica di aver avviato dal 2013 un processo di assunzione dei dipendenti di agenzie di recapito rimasti senza lavoro, di fatto con l'effetto di internalizzazione, parziale o totale, dell'attività di recapito, ma soprattutto di intervento sull'occupazione. senso: «a chiedere a Poste italiane SpA di fornire dettagliati elementi informativi in merito alla segnalazione della CONSOB, anche al fine di adeguarsi, se necessario, alle prescrizioni formulate nella medesima segnalazione». Sui punti 7) e 8) esprimo parere favorevole. esprimo parere favorevole. Vi sono poi i due ordini del giorno

degli uffici postali già presenti nei comuni rurali o nei comuni montani, secondo i principi del servizio universale definiti da Agcom». «a verificare che sia confermato il differimento dell'attuazione del nuovo piano di razionalizzazione di Poste italiane

prendiamo atto dei pareri relativi ai punti 4) e 5) della nostra mozione, dei quali chiediamo il voto per parti separate. Signor Sottosegretario, in ordine ai punti 1), 2) ed 8), lei ha proposto una riformulazione:

al termine del confronto in atto con gli enti locali, la lista completa degli uffici postali prossimi alla chiusura o interessati da una riduzione dell'orario di apertura, al fine di assicurare il rispetto degli obbilghi in capo al fornitore del servizio universale quale, in particolare, il mantenimento dell'operatività di un ufficio postale nel 96 per cento dei Comuni italiani;** senatore Arrigoni)*.

a sollecitare l'Agcom per lo svolgimento di una puntuale verifica di ogni misura di razionalizzazione degli uffici postali da parte di Poste italiane SpA, al fine di valutare di volta

il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dei 14 emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, adottati a Vienna nel 2005. Il testo in discussione reca anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno. È finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle previsioni del pacchetto di emendamenti alla Convenzione del 1980, derivanti dall'aggravarsi del contesto della sicurezza

delle materie nucleari, all'impiego generale delle materie e alla protezione delle installazioni, e con particolare attenzione al concetto di sabotaggio. La Convenzione del 1980 è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare, che fissa misure sulla prevenzione, la detenzione e le sanzioni delle violazioni in tale settore, con particolare riferimento alla fase del trasporto internazionale. In vigore a livello internazionale dal febbraio 1987, la Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 704 del 1982. Nello specifico gli emendamenti prevedono la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riferibili ad un uso non autorizzato e criminoso di detto materiale e dei relativi impianti. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Gli Stati parte della Convenzione sono altresì interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. È prevista inoltre la cooperazione tra i Paesi in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze, da realizzarsi in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi. I reati contemplati dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. Ulteriori aspetti sono relativi ai principi del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate. esecuzione consta, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, di dieci articoli, i primi due dei quali ineriscono all'autorizzazione alla ratifica ed all'ordine di esecuzione. Altre disposizioni relative ad ambiti di competenza degli affari esteri si rinvengono nell'articolo 3, che richiama alcune definizioni aggiuntive introdotte dagli emendamenti del 2005, al fine di chiarire in maniera univoca le accezioni utilizzate («protezione fisica attiva», «protezione fisica passiva», «piano di protezione fisica») e di individuare esattamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari. L'articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l'applicazione della Convenzione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile degli adempimenti internazionali, il Ministero dell'interno per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto, il Ministero dello sviluppo economico per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, il Ministero dell'ambiente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale, infine, per la formulazione di pareri tecnici, per gli accertamenti delle violazioni e per l'esercizio dei controlli sulla protezione. L'articolo 5 precisa le competenze per quanto attiene agli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, quale base necessaria per la predisposizione dei piani di protezione fisica passiva, mentre l'articolo 6 definisce il quadro autorizzativo per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché per i trasporti. Per tutti gli altri aspetti ed in particolare con riferimento alle sanzioni amministrative che il disegno di legge introduce, si rinvia alla relazione del collega della Commissione Giustizia. Si precisa Si precisa come dall'applicazione del provvedimento non deriveranno maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interessando la materia attività istituzionali già correntemente svolte a legislazione vigente da competenti amministrazioni. Da ultimo si evidenzia come l'accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

che riguardano proprio la tutela dei siti nucleari e, quindi, abbiamo anche previsto una sorta di nuovo strumento in grado di combattere questa condizione di eventuale aggressione e di messa in sicurezza introducendo una nuova fattispecie. Ai colleghi ricordo pure che per questo delitto di nuova fattispecie le competenze del tribunale sono in composizione collegiale.

quel disegno di legge, che adesso è alla valutazione della Camera, la fattispecie fosse meglio delineata. Per cui, abbiamo stralciato questa parte, per consentire alla Camera eventualmente di migliorare, rimanendo nel solco che ha tracciato il Senato. Questo è l'unico cambiamento che abbiamo apportato e si conferma la necessità di approvare il provvedimento al più presto, visto che abbiamo una scadenza internazionale a cui l'Italia deve arrivare preparata.